*relatore*. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2016 è la terza predisposta dal Governo Renzi. In linea con le precedenti, la Nota aggiorna le previsioni economiche di finanza pubblica contenute nel DEF presentato nel mese di aprile scorso in relazione alla maggiore stabilità e affidabilità delle informazioni disponibili sull'andamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica, e aggiorna gli obiettivi programmatici in considerazione delle raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'Unione europea. In allegato alla Nota di aggiornamento, il Governo ha trasmesso alle Camere anche la relazione al Parlamento, redatta ai sensi della con la quale si illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio periodo, si conferma l'impegno a ridurre il disavanzo e lo *stock* di debito delle amministrazioni pubbliche, si descrivono i presupposti dell'intervento, le linee generali e i contenuti della prossima legge di stabilità e dei suoi effetti sulla finanza pubblica e si descrive il nuovo piano di rientro verso il pareggio di bilancio in termini strutturali. I due documenti, da sottoporre all'approvazione delle risoluzioni parlamentari, illustrano pertanto la situazione macroeconomica e finanziaria che si è venuta a determinare nel corso dell'anno e le azioni che il Governo intende intraprendere nella prossima legge di stabilità per favorire la crescita economica del Paese nel rispetto degli obiettivi comunitari di stabilità della finanza pubblica e del raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio in termini strutturali. Il filo conduttore dei due documenti è la prosecuzione del percorso di bilancio dell'economia e dell'occupazione nel Paese intrapreso fin dall'insediamento del Governo. I primi due anni di Governo hanno prodotto risultati molto significativi. Il Paese è tornato a crescere dopo un lungo periodo di recessione e l'occupazione è tornata ad aumentare in modo permanente, come evidenziano anche gli ultimi dati diffusi dall'ISTAT. La crescita in Italia è tornata positiva nel 2014, ha accelerato nel 2015 e si sta rafforzando nel 2016. Le revisioni al rialzo recentemente operate dall'ISTAT sui dati annuali del PIL al 2014-2015 determinano a consuntivo un'evoluzione dell'economia italiana più positiva di quanto rilevato non solo in termini di prodotto, ma ancor più in termini di occupazione: 558.000 occupati in più ad agosto 2016 rispetto a febbraio 2014. Nell'anno in corso, nonostante la fragilità del contesto internazionale, dove si registra un generale rallentamento della crescita rispetto alle previsioni, l'economia italiana si mantiene in terreno positivo, anche se con un andamento leggermente inferiore rispetto alle previsioni di inizio anno. La crescita dovrebbe comunque attestarsi intorno allo 0,8 per cento su base annua. Il Governo, fin dal suo insediamento, ha perseguito una strategia orientata al rilancio degli investimenti sia pubblici che privati e in modo particolare al sostegno dei consumi interni attraverso l'aumento del reddito disponibile delle famiglie e la riduzione della pressione fiscale, fiscale, scesa dal 43,6 del 2013 al 42,1 del 2016. Questi fattori chiave, assieme all'ambizioso programma pluriennale di riforme strutturali, stanno contribuendo a migliorare la competitività del sistema produttivo. II pieno dispiegamento degli effetti delle riforme strutturali richiede un adeguato lasso di tempo ed è quindi indispensabile che la prosecuzione del percorso di consolidamento delle finanze pubbliche non sia di ostacolo alla definizione di politiche di bilancio orientate alla crescita. Ora si tratta di proseguire con convinzione su questo percorso virtuoso. Nella nota di aggiornamento, nella relazione al Parlamento e nella documentazione integrativa prodotta dal Ministro dell'economia messa a disposizione del parlamento e dell'UPB, il mix di interventi che il mix di interventi che l'Esecutivo si appresta a varare a partire dalla prossima manovra di bilancio sarà in grado di produrre una crescita programmata del PIL nel prossimo triennio pari rispettivamente a 1 punto percentuale nel 2017 1,3 punti percentuali nel 2018 e 1,2 punti percentuali nel 2019. Si è molto parlato in questi giorni proprio della validazione di queste cifre e del ruolo dell'Ufficio parlamentare di bilancio nell'esame dei numeri forniti dal Ministro dell'economia.

Credo che vada rivendicato con orgoglio questo passaggio dal Parlamento, che ha fermamente voluto la creazione e l'istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Questo nostro

È l'occasione per spiegare anche ai cittadini cosa sia l'Ufficio parlamentare di bilancio, che abbiamo voluto con la legge n. 243 del 2012, e che nient'altro è che un'autorità indipendente, un'autorità indipendente, non è certo un nuovo organismo superiore o laterale al Governo. Non abbiamo fatto una riforma costituzionale nottetempo. nemmeno di un organismo che trasporta a livello governativo, nei campi delle politiche fiscali ed economiche, le rigidità di un sistema paritario bicamerale.

di cui il Parlamento ha potuto godere nell'ambito delle ultime audizioni. A cosa servono queste stime? A creare un ulteriore inutile conflitto all'interno del dibattito? Certo che no. Servono a far sì che, di fronte a una previsione differente, si realizzi quella strana dicotomia, che qualcuno ha teorizzato, per cui se il Governo procede confermando le sue stime starebbe creando un muro contro muro con l'Ufficio del bilancio e se recede conformandosi starebbe procedendo a una sorta di resa incondizionata? Anche questo evidentemente non può essere. Si tratterebbe di un'inutile contraddizione creata da questo Parlamento. Con la creazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio abbiamo, invece, compiuto un atto di modernità per la nostra istituzione e per le nostre Camere. Ci siamo dotati di un'autorità indipendente che fornisce delle stime indipendenti. Quando le stime danno luogo a numeri sostanzialmente divergenti da quelli forniti dal Governo cosa bisogna fare? Lo dice la legge stessa: occorre risentire il Governo perché con quell'atto abbiamo semplicemente creato un punto di attenzione. Abbiamo, cioè, motivato una seconda audizione in cui approfondire i numeri che trovano un'opinione divergente nell'Ufficio parlamentare di bilancio.

Al primo livello si va a rivedere il quadro tendenziale. Ebbene, il quadro tendenziale rivisto dalla Nota di aggiornamento al DEF ci propone per il 2017 un PIL

Ciò significa forse che ci sono state delle divergenze nell'analisi con l'Ufficio parlamentare di bilancio? Non è così: diciamolo molto chiaramente. Questa prima e fondamentale stima è stata pienamente validata sia dall'Ufficio parlamentare di bilancio, sia da tutte le principali autorità

come tutte le autorità indipendenti e come l'Ufficio parlamentare di bilancio, sostiene che, a legislazione vigente, il PIL crescerebbe dello 0,6 per cento. Ecco allora che qui subentra la scelta fondamentale

la manovra, descritta per sommi capi nella Nota di aggiornamento, viene calcolata, prevista e stimata nei suoi impatti: si arriva così al quadro programmatico, che porta il Governo a dire che, a seguito degli esiti della manovra,

che vi è stata la divergenza e quindi abbiamo avuto l'opportunità di approfondire i dati forniti dal Governo. Faccio notare che, mentre le stime del quadro tendenziale si riferiscono a dati disponibili a tutti gli osservatori nella medesima modalità, le stime che portano al quadro programmatico, in maniera del tutto evidente, si riferiscono a dati che il Governo, in questa fase, detiene in maniera superiore, sia rispetto al Parlamento, sia rispetto alle altre autorità.

se questa divergenza fosse sostanziale e se fossero giustificate, alla fine, le stime del Governo. Possiamo dire che questo dibattito, per cui ringrazio tutti i colleghi che hanno preso parte alle sedute delle due Commissioni bilancio congiunte, ha dato modo al Governo di confermare, sia per analiticità, sia per convinzione e strategia, la bontà delle cifre che ci sono state proposte. Desidero sottolineare questo momento e salutarlo come un passaggio positivo per l'intero Parlamento, per la maggioranza e per le minoranze. Ora i nostri pareri potranno divergere sulla scelte che il Governo compie

relative agli immigrati e alle calamità naturali. È su questo che si dovrebbe concentrare il dibattito, ovvero sull'opportunità o no di compiere una scelta di politica economica di carattere espansivo, che non

Il prossimo anno potremmo quindi trovarci in un Paese più moderno, efficiente e competitivo e questo di per sé può rappresentare un moltiplicatore di fiducia per i cittadini e le imprese, in grado di spingere con nuova e maggiore forza la "nave Italia" verso lidi più tranquilli. La Nota di aggiornamento al nostro esame rappresenta pertanto una tappa fondamentale nel percorso descritto. I contenuti della Nota, adeguatamente integrati dal ministro Padoan, illustrano il quadro macroeconomico e di finanza pubblica che il Paese intende intraprendere per favorire la crescita. nello scenario tendenziale il PIL 2016, che scende dall'1,2 allo 0,8 per cento in relazione agli andamenti congiunturali della prima parte dell'anno, denota una fase di rallentamento della crescita economica. crescita economica. La constatazione che a livello internazionale e nazionale siamo di fronte a un rallentamento è la causa fondamentale delle scelte di politica economica che ci inducono a decisioni coraggiose di tipo espansivo, con l'obiettivo di andare a rafforzare la domanda interna, i consumi delle famiglie, gli investimenti, di migliorare le esportazioni.

Vorrei quindi soffermarmi su quel dato, che ho già voluto ricordare, dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni in rapporto al PIL, che sarà pari al 2,4 per cento per l'anno in corso, cento per il 2017, all'1,2 per cento per il 2018 e allo 0,2 per cento per il 2019. Rispetto al quadro, il rapporto *deficit*-PIL programmatico mostra dunque una traiettoria in discesa ma più graduale, in linea con l'intenzione del Governo di irrobustire la crescita, al fine di accelerare l'aumento dell'occupazione e di evitare che una *fiscal stance* eccessivamente penalizzante determini conseguenze negative sul tessuto sociale, già provato da anni di bassa crescita. Mi sembra che la vera natura della Nota di aggiornamento al DEF e della futura manovra risieda proprio in questo, ovvero nella volontà di percorrere quella via stretta, ma per noi fondamentale, che è l'unica che cerchi di tenere insieme la crescita, l'obiettivo di medio termine e il sostegno alle fragilità e anche quelle politiche redistributive che, al termine di un lungo periodo di crisi, diventano più che mai necessarie.

quindi di aumentare ulteriormente il *deficit*, o di avere una linea più conservativa che miri esclusivamente a tenere l'obiettivo di medio termine nei canali che ci eravamo dati.

pertanto sottolineato l'intendimento di conciliare stimolo alla crescita e rispetto delle pur stringenti regole fiscali;

recano in sé, prima di tutto, questo grande pregio. Non credo sia giusto dileggiare un Governo e una maggioranza che, numeri alla mano, portano al Paese proposte tese ad aumentare la fiducia. Certo, la fiducia è una cosa e i miraggi sono altro. Qui non vengono raccontati dei miraggi. Qui, con la tenacia di chi ha invertito il verso di un declino e sta lentamente ricostruendo una crescita, vengono prospettati degli scenari che nel medio periodo porteranno definitivamente il nostro Paese fuori dalla crisi. crisi. Come concordato con la Presidenza, lascerei questi scenari e questi numeri analitici agli atti, affinché possano essere colti anche in una futura lettura, anche perché questi giorni ci hanno consentito di mettere in evidenza gli aspetti più importanti e tutti gli elementi di crescita che, attraverso l'approvazione delle risoluzioni alla Nota di aggiornamento del DEF di oggi, intendiamo perseguire e che il Governo intende perseguire con noi. Ricordo che l'Annesso alla Nota di aggiornamento reca la relazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio periodo. Ai sensi del richiamato articolo 6, commi 3 e 5, la deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza l'aggiornamento del piano di rientro è adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Pertanto, l'esame del documento si concluderà con l'approvazione di due distinti atti di indirizzo: il primo, relativo alla relazione di cui all'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, da votare a maggioranza assoluta; il secondo, relativo alla Nota di aggiornamento da votare a maggioranza semplice. Le proposte di risoluzione ad entrambi i documenti dovranno essere presentate entro la fine della discussione. Dichiaro aperta la discussione. È iscritta a parlare la senatrice Bonfrisco. Ne

sarà un momento particolarmente difficile per il Paese, e quindi anche per il Governo. Dico questo perché adesso si dimostra sempre più ampio il divario tra le ipotesi o, meglio, le speranze di politica economica formulate dall'Esecutivo all'inizio dell'anno e, invece, i fatti che sono accaduti. Darei per acclarata la sopravvalutazione delle previsioni sulla crescita del PIL e sul miglioramento della finanza pubblica contenuta nel DEF della primavera scorsa e comprovata nella Nota di variazione che stiamo esaminando, perché di questo hanno già parlato tutti: osservatori, commentatori, addetti ai lavori. In questi ultimi quindici giorni tutti hanno avuto parole di perplessità e di particolare attenzione rispetto a un percorso economico finanziario svolto da questo Governo in quest'anno che solleva molti dubbi. Non credo ci sia nulla da aggiungere, anche per non smentire le note di ottimismo e di fiducia che dalla maggioranza

che non risultano nella realtà della nostra economia? Basti pensare al primo dato, quello sul quale veniamo poi giudicati da quelle regole europee che in tante occasioni abbiamo contestato. Il *deficit* di quest'anno,

Oppure, tanto per rimanere al *deficit*, a quello tendenziale del prossimo anno che, dall'1,4 per cento, diventa l'1,6 per cento. Oppure a quello programmato, che passa dall'1,8 per cento contrattato in sede europea al 2 Ma questa sempre maggiore distanza tra ipotesi e fatti non può non avere conseguenze; non resterà una mera discussione all'interno di questa o in altri consessi, dove le decisioni pesano ancora di più. Un persistente ottimismo non si limita ad aumentare gli effetti da minor crescita, un effetto già messo in evidenza dallo stesso Governo nel DEF di primavera; questo scarso realismo delle cifre mette in gioco l'attendibilità dell'Esecutivo, quindi, dell'intero Paese. Come dovrebbero reagire quegli operatori nazionali e internazionali che - vorrei

al Governo? Il quadro programmatico di finanza pubblica presentato nella Nota di aggiornamento non è pienamente significativo neanche sull'orizzonte annuale, essi dichiarano. D'altronde, i fatti hanno gioco facile sulle aspettative; quando queste assomigliano più a una immotivata speranza che a previsioni, diventano aleatorie, fondate su basi meno razionali. Mi chiedo: è ragionevole dubitare del modo in cui oggi la prevista rimodulazione delle imposte indirette (in altre parole la soppressione delle clausole di salvaguardia) si scarichi pressoché totalmente su quello 0,4 per cento, che è il tasso di crescita del PIL programmatico, rispetto a quello tendenziale del prossimo anno? La risposta è sì. L'economia, però, non è meccanica, non è: tolgo questo, aggiungo quello, ottengo quell'altro. Se si ripongono troppe aspettative sui modelli, si passa velocemente dalla dittatura dell'iperdato alla dittatura del non contemplato, quello che continuiamo a far finta di non vedere: un'evoluzione niente male! Allo stesso modo, perché tanta cautela da parte della Commissione sulle costanti richieste di spostare in avanti il pareggio strutturale? Non certo perché l'Europa valuta lo 0,1 per cento in più o in meno di crescita. Diciamolo chiaramente: dipende dal nostro debito pubblico, che non scende nemmeno in rapporto al PIL; anzi, aumenta, e come potrebbe essere diversamente con i livelli di spesa corrente primaria raggiunti e con una scarsissima crescita reale che non riesce a essere gonfiata opportunamente dall'inflazione? In questo documento programmatico il Governo preannuncia una manovra che, a dir suo, favorisce la crescita, articolata - per quanto è stato scritto e detto fino ad oggi ad oggi - sulla disattivazione delle clausole di salvaguardia, sull'anticipo pensionistico previsto dal recente accordo con i sindacati - meno male che è finita l'epoca della concertazione! - e su altre misure finalizzate alla riduzione del carico fiscale e contributivo delle imprese, all'aumento tanto agognato da tutti degli investimenti privati e della produttività, al miglioramento del mercato del lavoro e dell'occupazione, all'incremento degli investimenti pubblici e al sostegno al reddito delle famiglie. È un programma ambizioso? Certamente, ambiziosissimo. Ma, a parte l'entità della disattivazione delle clausole di salvaguardia, conosciamo quale sia la dimensione finanziaria vera dell'intero programma? A oggi, nonostante il perimetro delineato anche dall'ottimo intervento del collega Del Barba, tutto questo non appare chiaro. Tuttavia è possibile esprimere più di qualche riserva sui numeri che già leggiamo. Ad esempio, siamo proprio sicuri che l'anticipo pensionistico, la quattordicesima ai pensionati, la *no tax area* per gli *over* settantacinque, la ricongiunzione dei contributi previdenziali, la detassazione per chi attinge al fondo previdenziale pesino sulla collettività appena due miliardi annui? Sono tutti interventi che avrebbero il sostegno di chiunque, se i conti fossero fatti un po' meglio. Permetteteci di dubitare del fatto che l'INPS non si accollerà ulteriori oneri, come è già accaduto per gli esodati, perché non è nelle condizioni di farlo. Del resto, sul fronte copertura i dubbi non sono meno allarmanti, se essa è affidata, oltre che a un indiscutibile *deficit*, a una inafferrabile *spending review*, alla immancabile lotta all'evasione - della quale abbiamo già parlato molte volte - e a quell'apporto marginale della *voluntary disclosure*, il condono dei condoni sui condoni, che esprime una copertura che tutti auspichiamo e che poi, però, facciamo fatica a riscontrare. Anche quest'anno il Governo conta di far quadrare i propri conti grazie alla flessibilità che dice di ottenere da Bruxelles. Ma se questa è la qualità delle nostre previsioni, non meravigliamoci della diffidenza europea, nascosta dalle immancabili parole di circostanza, come quelle pronunciate recentemente dal commissario Moscovici, ma che tradiscono la realtà di ciò che si pensa di noi a Bruxelles. Diciamolo con onestà: la flessibilità ci è stata concessa, ma abbiamo mancato clamorosamente l'impegno che la giustificava già l'anno scorso. Abbiamo dimenticato le vicende dello scorso anno per ottenere l'autorizzazione a sforare? Il Presidente del Consiglio ha cambiato spesso motivazione: prima la clausola migranti, poi il pacchetto sicurezza e cultura, infine i costi della crisi libica, passando per la *querelle* sulla Turchia. Ma come sono state impiegate queste risorse? Cosa ha prodotto il rocambolesco cambio di linea difensiva? Nient'altro che *deficit*. In situazioni come queste, più flessibilità equivale inevitabilmente a più *deficit*, probabilmente lo stesso esito della prossima richiesta di sforare dello 0,4 per cento, basata sulle emergenze terremoto e migranti. Non meravigliamoci, quindi, se le nostre richieste vengono viste con molta circospezione, che non è solo da addebitare allo spirito burocratico delle istituzioni europee, del quale peraltro abbondano. Dovremmo renderci conto che giocare con i numeri significa anche giocare con le parole, un'attività che serve forse nelle vicende domestiche, quelle del Governo ovviamente, che ha bisogno di enormi programmi di spesa che diano l'impressione di dare tutto a a tutti, per gestire il consenso, per appianare i sempre più insanabili contrasti interni alla maggioranza o al partito di riferimento, per cercare di vincere la prossima scadenza referendaria e per altri più o meno evidenti interessi, che però non possono essere scritti in una manovra economico-finanziaria. Tutte cose legittime - si dirà - che appartengono alla democrazia. Ma gli interessi dei cittadini, delle famiglie, delle associazioni, delle imprese, gli interessi legittimi, sono assolutamente in secondo piano. Continuare sconsideratamente a fare scelte di politica economica basate sulla scarsa attendibilità delle previsioni è un po' come segare il ramo su cui è seduto l'intero Paese. E leggere i documenti ufficiali che le contengono è un po' come leggere, parafrasando Márquez, la cronaca di un disastro annunciato. E con questo, signor Presidente, nel completare il mio intervento

valorizzato i contributi che sono arrivati da molti (soprattutto all'interno della Commissione bilancio), non potrà che essere contrario. **Saluto

Signor Presidente, senatrici e senatori, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2016-2019 rispetto a quello contenuto nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile. Sottolineo questo aspetto, cioè il periodo di riferimento, a proposito della discussione che ha appassionato in questi giorni, perché le divergenze di proiezione dell'Ufficio parlamentare di bilancio rispetto al Governo vedono una differenza di previsione solo per il 2017 e solo per un aspetto, in un processo di validazione che peraltro è ancora aperto. Non mi soffermo sull'importante ruolo dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che credo sia davvero di supporto non tanto non tanto al Parlamento, quanto proprio al Governo, ma voglio solo sottolineare che il Governo attuale ha dimostrato in questi ultimi due anni una capacità previsionale molto più elevata dei Governi che si sono succeduti nell'ultimo decennio, i quali a consuntivo avevano differenze di previsione di vari punti, qualche volta addirittura di segno opposto. Però non voglio soffermarmi su questo aspetto, perché è già stato analizzato prima e

soffermare l'attenzione, nei pochi minuti che ho a disposizione, su alcune risposte del Governo alle raccomandazioni del Consiglio «Economia e finanza» dell'Unione Alcune mi stanno particolarmente a cuore: la raccomandazione n. 1 sulle regole di bilancio per le amministrazioni, sulle politiche fiscali locali e sul contrasto all'evasione e la raccomandazione n. 4 sulla lotta alla povertà. La raccomandazione n. 1 prevede, tra l'altro, il completamento della riforma del processo di bilancio nel corso del 2016 e di assicurare che la revisione della spesa ne costituisca parte integrante. il nostro quadro per le regole della finanza pubblica è stato completamente ridefinito in questi ultimi anni e ha permesso di rafforzare l'equilibrio sostanziale dei bilanci di supportare una puntuale programmazione degli investimenti. Ricordo solo che in questa revisione vi è stata anche l'approvazione delle modifiche alla legge n. del 2012, che comprendono, tra l'altro, l'inclusione nel saldo del Fondo pluriennale vincolato (strumento contabile che garantisce la copertura di spese imputate in esercizi successivi a quello in corso), che aiuta notevolmente la possibilità di programmare le attività degli enti locali. In questi giorni stiamo esprimendo il parere sull'Atto del Governo sui fabbisogni *standard*. poco vi sarà la chiusura nella legge di bilancio delle ultime annotazioni per i Comuni, affinché possano costruire, per la prima volta dopo tanti anni, il bilancio di previsione al Il nuovo quadro normativo di riferimento, delineando in modo chiaro, completo e coerente il concorso delle Regioni e degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica nazionali, pone le basi per una puntuale programmazione di medio e lungo periodo delle risorse sul territorio, che permette di rispettare gli equilibri di bilancio, da un lato, e favorire, dall'altro, il rilancio degli investimenti pubblici locali e il rispetto dei tempi medi di pagamento delle fatture commerciali su tutto il territorio nazionale. Veniamo alle altre attività che vengono messe in atto per rispondere alle raccomandazioni europee sulle politiche fiscali locali. La Nota di aggiornamento al DEF affida all'abolizione dell'imposta patrimoniale sulla prima casa rilevanti effetti di redistribuzione. Nel medesimo solco di interventi, il Governo afferma che valuterà con le prossime leggi di bilancio la possibilità di agire sull'IRPEF in base agli spazi finanziari disponibili. Nella valutazione complessiva della possibilità impositiva locale sugli immobili, diventa fondamentale la riforma del catasto.

previo allineamento delle basi-dati necessarie per valutare accuratamente gli effetti di gettito e redistributivi sui contribuenti, e distribuisce detto intervento tra il 2016 e il 2018. Veniamo a una considerazione importante, sulla quale però chiederei al Governo di riflettere: l'andamento del debito delle amministrazioni pubbliche per sottosettore.

a 2.220 miliardi di euro, le amministrazioni locali registrano una riduzione imponente di questo debito. Credo che di questo bisognerà tener conto. Il secondo aspetto che voglio sottolineare il contrasto all'evasione che ha registrato notevoli successi e ha rispettato esattamente le previsioni. Il gettito che si stima di realizzare nel 2016 è superiore a quello delle previsioni assestate di cassa. Le previsioni di incasso del 2016 sono superiori agli incassi registrati nel 2015 e il gettito permanente che si stima di realizzare nel 2016 è superiore al gettito permanente realizzato nel 2015. Aggiungo un'ultima battuta, una raccomandazione relativa alla lotta alla povertà e alla razionalizzazione della spesa sociale. Noi dobbiamo lavorare perché questo processo è buono, è avviato bene e il Piano nazionale di contrasto alla povertà è finanziato attraverso il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, con una dotazione di 600 milioni per il 2016 e di un miliardo a

la Nota di aggiornamento al DEF 2016, necessaria per adeguare le previsioni economiche di finanza pubblica al mutato quadro economico rispetto al DEF approvato ad aprile, non ci convince. Tutti i soggetti auditi dalle Commissioni bilancio di Camera e Senato - Banca d'Italia, Corte dei conti, ISTAT - hanno valutato le vostre previsioni come troppo fiduciose e ottimistiche. Addirittura l'Ufficio parlamentare di bilancio non ha validato il documento. L'intervento di ieri sera del ministro Padoan nelle Commissioni riunite non ha chiarito i dubbi e non ha dato risposta alle numerose osservazioni formulate. A mio avviso l'intervento del Ministro è stato sommario, deludente e avvilente.

le modalità di funzionamento dell'Aula e delle Commissioni sono state modificate e i lavori hanno avuto uno svolgimento inusuale inusuale e irrispettoso del lavoro del Parlamento. Questa mattina la Commissione bilancio è stata convocata con la modalità del messaggino - che purtroppo non ho visto - a seduta già iniziata, mentre in contemporanea erano in corso i lavori

Inoltre, Presidente, mi pare inaccettabile che argomenti di questa importanza come il DEF (credo che il DEF sia uno degli argomenti più importanti che vengono discussi in quest'Aula) possano avere uno spazio così ridotto: sette minuti per esprimere un giudizio su un documento in cui ci sono tutte le scelte più importanti per il Paese; è davvero assurdo, dato che a volte passiamo giornate intere, ore ed ore, a discutere inutilmente. veramente sconcertato dal senso che avete delle istituzioni e delle regole democratiche. Nel merito, le vostre previsioni sono, anche questa volta - per la decima volta consecutiva - inattendibili. Le misure attraverso le quali giustificate le previsioni di crescita sono inadeguate e i risultati saranno diversi da quelli previsti. Ma delle misure parleremo in occasione del Documento programmatico di bilancio 2017, quando verrà esaminato dall'Assemblea. Quello che mi preme sottolineare è che sbagliando le previsioni sul PIL si incrementa il debito pubblico che cresce in questo Paese in maniera inarrestabile, nonostante i proclami:

di dire basta ai proclami. Il ministro Padoan afferma: «Il debito comincia a ridursi nel 2017»; nel 2017, Presidente, il debito sarà più alto di oggi, se non altro per via degli interessi che saranno maturati, nonostante i tassi in ribasso. E sarà ancora più alto perché non si realizzerà il pareggio di bilancio e quindi il*deficit* maturato si aggiungerà al debito. del pareggio di bilancio al 2019, ma lo avete spostato di anno in anno. Che debito riducete, vice ministro Morando? Se non cresce il PIL, che rapporto riducete?

Disoccupazione drammatica, giovani senza lavoro in fuga all'estero (100.000 lo scorso anno), povertà dilagante, matrimoni azzerati (salvo quelli *gay*, che sono in crescita), nascita al minimo storico dal Dopoguerra in poi: dove state portando l'Italia? Possibile che non avete un briciolo di dignità per fermarvi un attimo a riflettere e raccogliere qualche suggerimento?

il pagamento dei 70 miliardi di euro di debiti della pubblica amministrazione alle aziende che li hanno maturati, che hanno fornito servizi, che hanno fatto lavori e che il Presidente del Consiglio si era impegnato a pagare il giorno di San Matteo (probabilmente non specificando l'anno)? Forse venti volte superiore Forse venti volte superiore ai 3,5 miliardi che stanziate per il rinnovo del contratto. Se invece di regalare gli 80 euro ai dipendenti pubblici prima delle europee aveste rinnovato il contratto dei dipendenti pubblici, fermo da otto anni, non sarebbe stato più giusto e logico? Visto che l'occupazione si crea solo riducendo gli oneri riflessi,

spero che non sia la versione definitiva. Credo che bisogna togliere l'elenco dei Comuni colpiti contenuto

Mandate i vostri tecnici, le vostre squadre, fate le vostre verifiche dei danni, ma non pensate di favorire qualcuno a danno degli altri. Lasciate alle Regioni di stabilire quali Comuni hanno subito danni e quali invece debbono

contribuire a questo dibattito con alcune considerazioni aggiuntive rispetto agli interventi che mi hanno preceduto, in particolare del relatore Del Barba e della collega Zanoni, che ringrazio. La Nota di aggiornamento al DEF 2016 giunge alla nostra attenzione in un momento estremamente delicato per la nostra economia che, dopo anni di recessione, ha ripreso a crescere, seppur in modo ancora insufficiente, a partire dal 2014. Gli scambi mondiali sono in piena gelata e la loro crescita per il 2016 si ferma ad oggi al 1,7 per cento rispetto alle stime di aprile che fissavano al 2,8 per cento; mentre per quest'anno, per la prima volta dal 2001, gli scambi cresceranno meno dell'economia che raggiungerà a livello mondiale un valore pari al 2,2 per cento. Questo dato relativo al crollo del commercio mondiale rappresenta uno dei principali fattori endogeni che danneggiano le prospettive di crescita della nostra economia, perché una crescita del commercio è sempre stata nella storia economica un segnale di forte espansione, soprattutto dei Paesi in via dì sviluppo che parallelamente si traduce in un forte aumento delle esportazioni verso questi Paesi da parte delle economie più avanzate. All'interno dell'economie avanzate, i più danneggiati dal crollo del commercio mondiale sono quei Paesi, come l'Italia, che sostengono la domanda aggregata attraverso le esportazioni, quale componente fondamentale del PIL. Negli anni della crisi la recessione è stata mitigata nel nostro Paese dalla capacità di esportazione che ha sfruttato la fase di crescita del commercio mondiale degli anni passati. Non è solo il commercio mondiale tra i fattori endogeni che penalizzano le nostre aspettative di crescita: anche la pericolosa spirale deflazionistica che sempre di più va ad adombrare l'economia nel suo complesso. Nonostante i massicci interventi monetari da parte delle principali banche centrali mondiali, Federal Reserve e BCE *in primis*, non si è riusciti a contrastare il fenomeno che, oltre ad agire sulle aspettative degli operatori economici con ricadute sul fronte della domanda, agisce negativamente sul fronte del rapporto reale tra *deficit* e PIL e tra debito pubblico e PIL. La caduta dei prezzi a livello mondiale non dipende, come da più parti sottolineato, dal calo del prezzo del petrolio, ma da fattori strutturali di più ampia portata. È di queste ore l'intervento del direttore del Fondo monetario internazionale, il quale ha affermato che la crescita media prevista a livello mondiale è troppo bassa e l'andamento negativo del commercio mondiale sarà ulteriore elemento di appesantimento. Il tema del rilancio degli investimenti a partire dai Paesi con un *surplus* commerciale e fiscale è necessario ed indispensabile per aiutare la crescita e gli investimenti pubblici e privati. In particolare, per l'Europa e l'area euro questi elementi sono urgenti. La bassa crescita acuisce gli squilibri e le ingiustizie della globalizzazione che solo con una crescita sostenuta consentono margini di riequilibrio. Di fronte a questo quadro congiunturale caratterizzato da potenti fattori endogeni le politiche messe in campo dal Governo in questi anni sono state un forte fattore di attenuazione dei loro effetti negativi garantendo una crescita del PIL anche senza il concorso di quei fattori che storicamente hanno salvato la nostra economia, come una incontrollata spesa pubblica e il commercio estero. pertanto credibili le previsioni del MEF e del nostro Ministro dell'economia. Di fronte a questo quadro, voglio portare alla vostra attenzione quattro fattori che ritengo fondamentali: mesi di crescita consecutiva, il mercato dell'auto ha improvvisamente frenato a luglio, segnando un -1,8 per cento, con ricadute sulle previsioni di crescita del Ma secondo i dati diffusi a fine settembre, ad agosto tale mercato ha segnato un incremento pari al 9,5 per cento, recuperando ampiamente il dato negativo di luglio, un dato che si manterrà positivo anche a fronte della previsione di un nuovo calo a settembre.

La stessa produzione industriale vede un miglioramento diffuso nel manifatturiero in nove settori su quindici presi ad esame. La capacità di traino del settore manifatturiero è centrale per il nostro Paese. Gli interventi volti a sostenere l'ammodernamento dei macchinari industriali hanno dato risultati molto positivi attraverso il superammortamento e la cosiddetta legge Sabatini, consentendo di migliorare la nostra competitività e la nostra produttività, spingendo peraltro la produzione in un settore come quello dei macchinari industriali in cui siamo *leader* a livello mondiale. Siamo nella fase della quarta rivoluzione industriale e l'impegno attraverso il Piano nazionale industria 4.0 ha carattere strategico per essere al passo con le economie più avanzate.

del PIL mondiale. Abbiamo quindi un patrimonio irrinunciabile da sostenere. Passo al secondo fattore. Sul piano degli investimenti, dopo il crollo degli anni della crisi, il Paese ha ripreso a crescere e finalmente dal 2017 avremo il segno «+» sulle risorse investite in infrastrutture e opere pubbliche. Non solo la pianificazione sulle grandi opere dei tre anni precedenti si tradurrà in risorse effettivamente investite per opere che si completano, ma anche gli investimenti delle Ferrovie dello Stato, dell'ANAS, del comparto idrogeologico e delle piccole e medie opere pubbliche dei Comuni, grazie al superamento del Patto di stabilità, iniziano a incidere in modo concreto sul livello dei nostri investimenti, con ricadute sull'economia reale. Il *bonus* per le ristrutturazioni edilizie, l'efficientamento energetico e il loro ampliamento per il 2017 aumenteranno l'importante volume di investimenti generati, che ammonta già a 28 miliardi di euro. Nel settore del turismo e dei servizi in generale l'aumento dei flussi turistici e del volume di ricchezza generato segna passi molto significativi in termini di ricchezza prodotta.

Dobbiamo concentrare le risorse disponibili perché il nostro sistema industriale, in particolare quello manifatturiero, possa, attraverso lo sfruttamento del Piano nazionale industria 4.0, essere al passo con le economie avanzate. Dobbiamo naturalmente anche intervenire con misure che aiutino a produrre politiche di riequilibrio e giustizia sociale. Da questo punto di vista, la messa in campo di strumenti come il reddito di inclusione sociale un primo segnale annunciato sul sostegno alle famiglie con figli a carico rappresentano, a mio avviso, un altro elemento che si va a integrare agli altri che sono già stati indicati nelle relazioni

eccellenze e centri di servizi e infrastrutture di valore nazionale al Sud, che rappresenta per questo Paese un'opportunità di crescita sostenuta a due cifre e per lungo tempo.

Signor Presidente, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza contiene innegabilmente dati molto negativi

nel corso dell'anno si sono fatte delle previsioni assolutamente sbagliate, scorrette e troppo ottimistiche, ma anche un altro fattore nuovo, ossia un un aggiornamento che prevede dei numeri ancora troppo ottimistici. Questo non lo diciamo noi, ma l'Ufficio parlamentare di bilancio che, come tutti sappiamo, non è d'accordo con i contenuti principali della Nota di aggiornamento preoccupa tutti noi. Allo stesso modo, ci preoccupano le valutazioni della Banca d'Italia. Il Governo ha deciso di ignorare i richiami dell'Ufficio parlamentare di bilancio e della Banca d'Italia e di proseguire con un aggiornamento

che determinerà il futuro e la sopravvivenza di questo Governo. Il Governo ha bisogno di affrontare la fase referendaria con ottimismo e dei dati falsi pur di raggiungere un obiettivo che gli sta a cuore, ovvero superare indenne la prova del 4 dicembre

Anche il ministro Padoan prevede una crescita sicuramente al di sopra delle realistiche possibilità del nostro Paese

che era ed è necessaria. Questi 19 miliardi di flessibilità sono purtroppo stati bruciati per l'unico obiettivo di cercare un facile consenso. È un dato che ci preoccupa, anche perché è evidente a tutti che questa flessibilità non potrà essere concessa all'infinito all'Italia. Il fatto che il Governo Renzi abbia avuto tali opportunità al di sopra di qualsiasi altro Governo precedente evidenzia il fallimento delle politiche economiche di questo Governo. È evidente che i dati che il presidente Renzi e il Governo ci propongono sono assolutamente fuori dalla realtà: non c'è crescita non c'è crescita ed è così non perché il contesto internazionale ci impedisce che tale crescita si possa avviare. Si sono trovate delle scuse rispetto a questa mancanza di crescita che sono assolutamente risibili. Si è detto che uno dei motivi per cui non c'è crescita è la Brexit. Non c'entra niente con ciò che sta accadendo nel nostro Paese, come non c'entra alcunché l'esito incerto del voto negli Stati Uniti. Queste sono le argomentazioni che portate rispetto ad un'Italia che arranca e non riesce a crescere.

nel 2017, quando finiranno le norme sulla decontribuzione sulle nuove assunzioni, la disoccupazione avrà una nuova crescita. C'è la fuga di giovani: è stato detto che l'anno scorso più di 110.000 giovani sono fuggiti dall'Italia. Noi importiamo immigrati ed esportiamo giovani laureati che cercano di fare fortuna. È un Paese ormai allo sbando. È una follia quella che stiamo vivendo.

La diminuzione della spesa pubblica è attuata solo sulle spalle degli enti locali e sull'impegno dei sindaci e delle Regioni e con una spesa centrale che aumenta ancora di più.

La realtà è diversa: è quella di un Paese che arranca, fa fatica, con i cittadini che soffrono una situazione drammatica. Purtroppo, la realtà è che i vostri conti sono truccati, irrealistici e non porteranno alla salvezza della nostra economia.

considerazioni assumono del tutto il quadro rappresentato dalla Nota di aggiornamento al DEF e quindi, sostanzialmente, un peggioramento delle prospettive di crescita della nostra economia. Naturalmente sono diversificate e contrapposte le interpretazioni sul fenomeno e le valutazioni sulle misure messe in atto, ma a mio giudizio il Governo fa assolutamente bene a rafforzare le scelte per la crescita e lo sviluppo, sebbene in un contesto di sostanziale rispetto della traiettoria di equilibrio della finanza pubblica e nel rispetto tendenziale

ma certamente vanno messe in campo, perché la crisi di questi anni e la difficoltà ad uscirne colpisce in modo duro le fasce più deboli della nostra popolazione, allarga le diseguaglianze tra strati sociali e tra generazioni: è questa la nostra preoccupazione. Credo che la risposta stia anche in un *welfare* inclusivo e proattivo. A mio giudizio vanno in questa direzione provvedimenti che abbiamo sentito citare solo in un paio di interventi, che sono già parte consolidata del nostro ordinamento.

Penso che la sanità pubblica sia stata, almeno in questi anni, sicuramente un laboratorio di rigore e innovazione.

nella prossima legge di bilancio dobbiamo assolutamente onorare, con finanziamenti adeguati, le sfide dei LEA, le sfide dei farmaci innovativi e il personale, perché se in questo periodo di crisi le prime vittime sono state i cittadini, che hanno visto oggettivamente contrarsi l'offerta dei servizi, le seconde vittime sono tutti gli operatori, che hanno retto in un contesto difficilissimo il servizio.

Signor Presidente, signor vice ministro Morando, non credo di essere da premio Nobel se le dico che l'Italia, a differenza degli altri Paesi europei, sta uscendo solo ora dalla lunga crisi

non hanno pagato. È stata imposta al Paese una cura draconiana che ha notevolmente peggiorato la situazione economica e sociale, contribuendo solo in misura modesta al miglioramento dei conti L'interrogativo se non era il caso di seguire l'esempio francese, spagnolo o finlandese (per citare solo tre Stati che non hanno rispettato i parametri europei), ovviamente rimane senza risposta. Il Presidente della Repubblica del tempo e i presidenti del Consiglio Monti e Letta invece ci hanno voluto portare verso questa austerità merkeliana.

il suo dovere, quindi la base di partenza per il 2017 e gli anni successivi è più solida che non negli anni precedenti, ma non scevra da

pur nel rispetto delle regole fondamentali dell'Unione europea, che ci sia la flessibilità per l'immigrazione e per il terremoto che l'Italia è costretta ad affrontare. Soprattutto, però, signor Vice Ministro, noi crediamo che con il suo

Signor Presidente, ci troviamo ad operare in un contesto di ripresa globale molto lenta e di decelerazione della produttività del lavoro, che sono in gran parte il riflesso di un rallentamento del processo di accumulazione. Dall'altro lato vediamo che la nostra finanza pubblica si muove in un contesto molto stretto, per quanto stiamo cercando di conquistare margini di flessibilità in ambito europeo. In questo contesto, è assolutamente necessario che la legge di bilancio stabilisca delle priorità molto precise e dia stabilità e programmi per incidere sulle aspettative alcuni interventi che, secondo me e altri, sarebbero necessari. Innanzitutto, sarebbe controproducente disseminare pochi soldi su molti obiettivi con strumenti di breve o brevissimo orizzonte. Bisogna, al contrario, concentrare il proprio sforzo sugli investimenti e, in particolare, su quelli in più in grado di creare la domanda. Il problema che abbiamo non è tanto di costo del lavoro ma di domanda. È su quella che occorre intervenire, e gli investimenti più efficaci

Il sostegno agli investimenti privati va pure esso sostenuto, ma poiché, come ci ricorda la Nota di accompagnamento, quelli in macchinari e attrezzature non hanno mostrato l'abbrivo atteso, è importante concentrare le risorse per favorire interventi di tipo selettivo, per sostenere gli investimenti

Bianco, è che la legge di bilancio non introduca riduzioni al finanziamento pubblico di parte corrente del Servizio sanitario nazionale rispetto al quadro tendenziale previsto nella Nota di aggiornamento del DEF. Non possiamo operare tagli su questo. L'Ufficio parlamentare di bilancio ci ricordava in una precedente nota che le persone che rinunciano alle cure per motivi economici sono passate dal 3,6 per cento del 2004 al 6 per cento nel 2013, e questa cifra è più alta se consideriamo le fasce più povere. Quindi noi, per garantire i nuovi LEA ed evitare razionamenti che derivano, ad esempio, dalle distanze da percorrere e dalle liste d'attesa, L'ultimo punto che vorrei toccare riguarda la strategia, evocata, del contrasto all'evasione. Un aspetto su cui non si concentra abbastanza l'attenzione è che le imposte dichiarate, fuori quindi dal rischio di accertamento, ma non versate, stanno aumentando moltissimo: a 15,8 miliardi di euro nel 2013. Noi non dobbiamo assolutamente - come si legge sui giornali - rispondere a questo fenomeno

non solo per quanto riguarda il proprio debito fiscale ma anche il fisco che si raccoglie dagli altri: quindi anche l'IVA e le ritenute sul lavoro. Questo fenomeno sta crescendo:

preluda a un'emersione del contante, perché questo veramente espone, qualunque sia il paletto che vogliamo mettere (a meno che non sia un paletto che elimina il problema alla radice) al grosso rischio di tradursi in una grossa operazione di riciclaggio legale di denaro sporco. L'ultimo aspetto che vorrei sottolineare sull'evasione fiscale è che bisogna che nella legge di bilancio, visto che non lo si è fatto con altri strumenti fino ad ora, si prevenga la paralisi operativa in cui si troverebbe ad operare l'Agenzia delle entrate quando il 31 dicembre scadranno per legge gli incarichi dirigenziali attribuiti in via transitoria, con una norma che abbiamo introdotto nella legge di bilancio dell'anno scorso per iniziativa parlamentare. Mi aspetto che su questo il Governo abbia messo a punto in un anno una strategia strategia che diventa sempre più urgente, anche a seguito dell'inibizione ai concorsi che è avvenuta dalle recenti pronunce, peraltro contraddittorie l'una rispetto all'altra, del Consiglio di Stato. Questi sono gli aspetti che considero prioritari per la legge di bilancio, e insieme a me tanti altri senatori.

Vi ricordo che quella era una favola che si raccontava ai bambini; questa è realtà, purtroppo. Arrivo al sodo. Non voglio nemmeno commentare quanto hanno detto su questo DEF coloro che non sono vostri nemici (facciamola passare così): Banca d'Italia, Corte dei conti, Istat. Non lo commento neppure, perché credo che chi ama le cose vere non ha bisogno di queste affermazioni. affermazioni. Parlate di favorire la crescita e di lotta alla povertà. Vi do alcuni dati, e voi siete al Governo da due anni e mezzo: 1,470 milioni di famiglie in condizioni di povertà assoluta,

e sta comportando per il Sud uno spopolamento senza precedenti. Lo dico da troppo tempo, e voi fate finta di non accorgervene.

Voglio ricordare che avete regalato 20 miliardi di euro ai padroni senza un minimo di occupazione; l'unica cosa che quella norma ha prodotto (anche questi dati vengono da

perché nessuno lo assumerà; non avrà nessun diritto, se non quello, forse, garantito dall'Inail. Però anche di questo non si parla, o non ne volete parlare. Quello che interessa a voi è eliminare i diritti che la nostra Costituzione ci garantisce, ancora per un po', e che spero continuerà a garantirci, perché sono sicuro che i cittadini e le persone hanno capito chi siete e cosa volete fare.

In sette minuti non si può dire tanto, ma quando parlate di investimenti io sul serio faccio fatica anche a seguirvi da questo punto di vista.

si è tolto ogni vincolo alle imprese, le quali ormai non hanno alcun vincolo; e, come ho detto prima, questo non ha prodotto alcun beneficio per i lavoratori. Quindi siete partiti dalla cancellazione dei diritti e dai *voucher* (come ho detto prima) per arrivare ai buoni pasto. Lo dico in modo provocatorio: non vorrei che in questi giorni si parlasse anche di stipendio virtuale, perché è l'unica cosa che ancora non avete fatto. Dopodiché i lavoratori li avete massacrati: non hanno più alcun diritto e voi continuate a parlare di crescita e di lotta alla povertà.

riguardante il reddito minimo garantito, che c'è in tutta Europa (in tutta Europa, visto che parliamo sempre di Europa quando vi fa comodo). Bene, voi vi presentate con una (non so come altro definirla), quando, a detta dei migliori analisti ed esperti di questo campo, per avere una lotta vera alla povertà il Governo dovrebbe investire 7-8 miliardi di euro all'anno. Allora io mi domando e domando a voi: come mai si regalano 20 miliardi di euro e non si crea alcuna occupazione (e voi siete consapevoli di questo), quando bisogna veramente aiutare le persone e le famiglie in difficoltà, ve ne venite sempre con delle cose che sono una miseria e che non rendono alcuna dignità alle persone? Sarete responsabili di questo disastro, soprattutto quelli che hanno fatto una campagna elettorale dove c'erano otto punti ben precisi, dei quali non è rimasto nulla. i vostri alleati di destra (anche se non so più definire chi è di destra e chi è di sinistra in mezzo a voi) dicono apertamente che voi state adottando le politiche del loro Governo. Io sono convinto e sono certo che le persone perbene (perché questo Paese è composto da persone perbene) non ve lo perdoneranno. Signor Presidente, fin dalla premessa nel DEF il Governo pone l'accento sulle ricadute positive, secondo lo stesso Governo, nel medio termine della riforma cosiddetta della buona scuola. La La scuola rappresenta di fatto la più grande azienda del Paese: abbiamo 8.384 istituzioni scolastiche, più di 41.000 sedi, più di 700.000 docenti, cui deve essere aggiunto il personale amministrativo, dirigente e ATA. Tuttavia, l'abbondanza di risorse promesse e sbandierate dal Governo e dalla maggioranza viene di fatto smentita dai documenti che analizzano la spesa dello Stato. Leggendo i dati contenuti nella relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2015, si evince che le risorse per il comparto non sono aumentate, anzi, al netto delle spese per le assunzioni, i fondi a disposizione restano praticamente identici a quelli relativi relativi all'anno finanziario 2013. Gli 800 milioni di euro stanziati non sono sufficienti; infatti, non sarebbero neppure sufficienti a coprire il salario minimo per adeguare le buste paga all'inflazione. Abbiamo quindi una classe di insegnanti che che rimane la meno pagata d'Europa. Il piano assunzionale straordinario per gli anni 2016-2017 aveva poi lo scopo dichiarato di finirla per sempre con gli organici scoperti e gli incarichi di supplenza annuale, oltre che a rimediare ai contratti a termine, sanzionati dalla Corte europea. Tuttavia apprendiamo da uno dei portali più seguiti dalla scuola - il portale di Orizzonte scuola scuola - che ci sono ancora 10.500 posti vacanti sui 63.712 messi a bando per il triennio. In sintesi, la situazione è tutt'altro che risolta e a questo si aggiunge il caos del concorsone e della mobilità.

sarebbe opportuno fermarsi per un'attenta valutazione degli effetti da questa prodotti sulla qualità del servizio e le condizioni di lavoro di dirigenti, docenti e personale ATA. Infatti, l'anno scolastico è iniziato nel peggiore dei modi, con disfunzionalità e e iniquità. Basti pensare alle molte classi ancora scoperte a causa dei ritardi e dei gravi errori commessi dall'amministrazione nella gestione delle operazioni di mobilità e nelle assunzioni dei supplenti. Il primo anno di sperimentazione dell'obbligo dell'alternanza scuola-lavoro, poi, non ha dato esiti migliori e i frutti sperati non sono arrivati. Sorvolo sulla questione della finta abolizione delle Province e su tutto il caos che si è ingenerato nel passaggio di competenze alle Città metropolitane e alle Regioni. L'edilizia scolastica non sta messa meglio. Ieri sera il *premier* a «Politics» ha addirittura dichiarato che il suo Governo ha stanziato più soldi di tutti, che è una affermazione non totalmente corrispondente al vero, considerato che molti dei fondi stanziati non afferiscono al Governo Renzi ma a prestiti della BEI e a fondi già stanziati da Governi precedenti. Ha abbozzato solo qualche scusa sulla carenza di controlli e problemi di burocrazia per i tetti che ancora crollano. L'università e la ricerca non stanno messe meglio, siamo ancora molto indietro: siamo al 27° posto per gli investimenti in ricerca e al 35° posto per numero di ricercatori. Il comparto AFAM, dopo tre anni di stallo in Commissione e due anni di cantiere AFAM, solo in questi giorni ha visto venire alla luce un testo unificato e non si sa quale quale sarà la sorte. che rischia di mettere in paralisi e non stabilizzare molti ricercatori a tempo determinato in enti di ricerca fondamentali, quali ENEA, ad esempio.

In materia di cultura vorrei concludere con due osservazioni di attualità. Infatti nel DEF non c'è traccia del collegato Atto Senato 2287 recante «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo», approvato in prima lettura al Senato il 6 ottobre 2016. Lo stesso silenzio è riservato allo spettacolo dal vivo; dal vivo; negli ultimi anni abbiamo assistito a una trasformazione del comparto in un'impresa commerciale legata a logiche di mercato e ad algoritmi sterili. sterili. Pensiamo che, per quanto riguarda scuola, università, ricerca scientifica e cultura, nel DEF sia elencato un libro un libro dei sogni di quello che il Governo avrebbe voluto fare e di quello che forse il Governo farà. Noi rimaniamo in paziente attesa degli investimenti che da anni chiediamo siano fatti in questi tre comparti. È di attualità quindi vogliamo battere sugli investimenti necessari per l'università

Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, i chiarimenti forniti ieri sera dal ministro Padoan alle Commissioni riunite, rivelano che siamo di fronte ad una manovra in linea con quelle precedenti, ma che genera ancora più *deficit*. Eppure eravamo rimasti alle parole del *premier* Renzi di lunedì scorso, secondo cui l'azione del suo Governo non si baserebbe sui *bonus*, ma su misure strutturali. Per misura strutturale si intende quella che non è occasionale o congiunturale e che possiede una solida copertura finanziaria. Le principali azioni intraprese in questi tre anni non hanno la prima caratteristica. Eppure, laddove abbiano la prima proprietà, si basano largamente su coperture assicurate da clausole di salvaguardia su IVA e accise. La legge di bilancio per il prossimo anno sarà al 60 per cento costituita da misure volte a coprire la clausola rimasta attiva per il 2017, che vale 15 miliardi, coperta con 13,3 miliardi di *deficit*. Quindi è il Governo dei *bonus*, ma anche delle clausole. Accanto alle clausole di salvaguardia, che rimarranno comunque in eredità alle manovre successive (lo ricordiamo per memoria: 20 miliardi e mezzo per ciascuno degli anni 2018 e 2019) ci sono le clausole di flessibilità. Questo costituisce l'altro grande imbroglio della politica economica del Governo. Infatti la gente è convinta che l'Europa, autorizzando la clausola di flessibilità sui migranti, mandi soldi all'Italia per coprire le spese legate alla loro permanenza nel Paese, in attesa del vaglio delle domande per un eventuale asilo. In realtà, significa che la Commissione europea autorizza il nostro Paese ad una ulteriore spesa in *deficit* per 3,3 miliardi, per la quale l'Italia dovrà emettere ulteriori titoli di debito pubblico. per affrontare la crisi dei migranti l'Italia ha ricevuto dalla UE solo 112 milioni nel 2016, quindi l'accoglienza dei migranti oggi la paghiamo noi, ma la pagheranno i nostri figli e sicuramente anche i nostri nipoti, considerato che ormai l'Italia emette buoni del Tesoro di durata cinquantennale. La valutazione che diamo di questo sesto documento previsionale del Governo Renzi può essere fatta sul raffronto con le previsioni mancate dal 2014 ad oggi. L'azzeramento del livello dell'indebitamento netto, che secondo le previsioni del 2014 avrebbe dovuto raggiungersi a ridosso del 2017, ora si sposta a data da destinarsi, cioè ben oltre l'orizzonte programmatico del 2019. Oltretutto, va sottolineato che la spesa per la ricostruzione post-terremoto (per la quale si è chiesta una ulteriore clausola di flessibilità dello 0,2) è da considerare una spesa davvero eccezionale, perché rappresenta il giusto risarcimento per i superstiti superstiti del sisma del centro Italia e un investimento nel patrimonio abitativo e pubblico delle zone colpite che muoverà sicuramente l'economia di quelle zone. Al contrario, per i migranti, si tratta di risorse pubbliche utilizzate male per un evento largamente previsto e quindi evitabile. La spesa per la gestione dei migranti si è quasi triplicata in questi ultimi anni. L'importo previsto per il 2017 sarà pari a quello dello scorso anno, cioè di 3 miliardi e 300 milioni. Quindi nulla di imprevisto, ma piuttosto il risultato di una pessima politica estera che non ha fatto valere l'Italia sui tavoli europei. Con la nuova spesa in *deficit* si sposta, di conseguenza, anche il traguardo verso la riduzione del rapporto debito - PIL, che rimane nel 2017 stabilmente sopra il 132 per cento, anche nel nuovo quadro programmatico. Lontanissimo, ovviamente, il livello del 120 per cento considerato "sostenibile" per i conti pubblici italiani, che pure era stato assicurato come obiettivo raggiungibile per il 2018 nel DEF di due anni fa. Intanto, il Governo continua, e va sottolineato, a beneficiare del regalo di Mario Draghi e della BCE, che continuerà ad acquistare i nostri titoli almeno fino a tutto il prossimo anno. Vorrei aggiungere un'altra considerazione: penso che un documento economico e programmatico dovrebbe contenere valutazioni serie sulla sostenibilità del debito. Infatti parte della manovra per il prossimo anno verrà sostenuta grazie ai minori interessi passivi preventivati per quasi 5 miliardi. Le stime del prodotto interno lordo scendono rispetto al quadro programmatico d'inizio mandato, nonostante un crescente livello della spesa pubblica posta dal Governo a presidio della crescita del PIL. 28,5 miliardi di crescita del PIL nominale nel 2017 sembrano ora poco realistici, perché si è in presenza di un livello di inflazione prossimo allo zero. Ma il problema non è quanto siano accurate le previsioni sull'incremento del prodotto interno lordo, che cresce nonostante l'azione largamente depressiva del Governo. La domanda a cui bisogna rispondere è per quale ragione gli investitori scappino dall'Italia. Infatti, sia il risparmio italiano che il denaro degli investitori mondiali, purtroppo, non sono attratti dalle attività produttive del nostro Paese. La nuova manovra quindi, si baserà su misure *una tantum*, sui tanti, troppi, *bonus* e sui pochi tagli agli sprechi. Continuiamo a leggere una pericolosissima sottovalutazione delle dinamiche della spesa corrente. Quello che manca nella Nota sono proprio le proposte; prima fra tutte, come fare uscire da sotto il mattone il risparmio dei nostri concittadini, e quindi come ricreare fiducia nel sistema Paese. Al calo del reddito delle famiglie italiane si deve rispondere con politiche che garantiscano una tenuta duratura del potere di acquisto. Per questo servono fatti concreti. nonostante il racconto renziano, le cronache italiane parlano ancora di furbetti del cartellino, di scuole senza professori a un mese dall'inizio dell'anno scolastico, di soffitti che crollano nelle classi, di finti profughi che costano agli italiani 35 euro al giorno, di degrado urbano, di casi di corruzione, di morti in corsie d'ospedale: cioè di una Italia che non ha assolutamente cambiato verso. Allora diventa anche inutile spostare il dibattito sul merito dei 47 articoli modificati della Carta fondamentale. Il no al *referendum* deve essere un chiaro voto contro la politica economica disastrosa di questi anni del Governo Renzi, che ha indebitato il Paese a un livello *record* e che continuerebbe qualora il Paese, a dicembre desse, la fiducia a questo Esecutivo. Alla luce di quanto evidenziato, per Forza Italia sarebbe stato opportuno valutare di proporre non una risoluzione alla Nota di aggiornamento al DEF - come abbiamo fatto - ma una mozione di sfiducia al Governo.

Come è stato detto, la Nota disegna un quadro di riferimento macroeconomico per una legge di bilancio che si muove e si muoverà lungo un sentiero stretto, che è delimitato, da un lato, da andamenti del quadro economico europeo internazionale che non sono rassicuranti (c'è una ripresa, ma è in deciso rallentamento) e, dall'altro, da paletti che continuano a essere assai rigidi e che sono imposti tutt'ora dalle regole europee.

come già l'arresto della crescita nel secondo trimestre ha segnalato, a causa di debolezze strutturali esistenti che conosciamo molto bene e che dobbiamo continuare ad aggredire con riforme che sono state solo in parte avviate e che necessitano ancora di numerosi interventi. Poi ci sono i paletti dell'Europa. Noi ci siamo impegnati, per godere della flessibilità lo scorso anno e per quest'anno, ad un *deficit* di bilancio nel 2017 pari all'1,8 per cento rispetto al 2,4 che è previsto per il 2016. Ma il quadro macroeconomico è cambiato: quindi, alla luce di questo rallentamento, rispettare oggi quell'impegno significherebbe una manovra prociclica fortemente restrittiva che penalizzerebbe fortemente la già modesta crescita in atto e la frenerebbe intorno allo 0,5-0,6 Questo è esattamente il contrario di ciò che un buon manuale di macroeconomia ci suggerirebbe di fare, perché quello che serve in realtà in questa fase sono interventi anticiclici. Credo che Credo che la politica di bilancio contenuta nella Nota di aggiornamento proponga esattamente un intervento di questo genere che porta il *deficit* dall'1,6 per cento, a politiche invariate, al 2 Quindi, in qualche modo sfrutta uno spazio fiscale disponibile che è stretto, come ho detto, sia a livello domestico, dato il rallentamento in atto, sia a livello europeo, viste le regole certamente criticabili, ma che tutt'ora esistono. Nel valutare l'impatto di questa manovra, sono state avanzate dall'Ufficio parlamentare di bilancio delle obiezioni. Si è detto che, a fronte del 2 per cento di *deficit*, era troppo ottimistico

Come sappiamo, questo è stato fatto sulla base di una stima media di *consensus* tra vari modelli di previsioni utilizzati. Credo dunque che sia importante ribadire che non è sulla necessità e sulla natura anticiclica della manovra

Si può dire che questa sia una differenza più di forma che di sostanza e nasce ovviamente dalla eterogeneità dei metodi e dei modelli utilizzati per le analisi e le stime, che non deve sorprendere perché è riconducibile a quell'eclettismo e a quel pluralismo che oggi contraddistingue la scienza economica, teorica e applicata.

ed abbiamo sempre ritenuto fondamentale questo ruolo e questa autonomia), ma perché bisogna anche assegnare un corretto significato alla lettura e all'utilizzo delle analisi e delle previsioni che l'Ufficio A tale riguardo è importante anche sottolineare, per tornare alla Nota di aggiornamento, che le misure d'intervento in essa contenute sono giudicate da alcuni troppo deboli, non in grado di stimolare effettivamente l'economia. Qui bisogna intendersi. Ovviamente si può sempre dire che si può fare di più e meglio, però mi sembra che da parte di alcuni venga avanzata la proposta di violare apertamente e unilateralmente le regole dell'Europa: fare di più andando

lo scenario che si sta profilando per l'anno prossimo: ricordiamoci che nel marzo del prossimo anno scade, almeno ufficialmente, la politica monetaria non convenzionale della BCE, e non è affatto scontato che questa politica possa continuare nelle modalità e nella quantità fino ad oggi realizzata. Mi chiedo allora se per l'Italia sia avveduto, in uno scenario di questo genere,

che verrebbe dal fatto di dover pagare sicuramente dei tassi di interesse assai più elevati. Concludo ritenendo che sia importante ribadire che la manovra nella Nota di aggiornamento cerca di utilizzare a fini anticiclici degli spazi potenziali disponibili, ma ribadendo, all'interno di un contesto europeo e di un'area dell'euro, dell'euro, certe regole che abbiamo criticato e continuiamo a criticare, e che vorremmo cercare di cambiare. Ma queste regole in realtà sono fondamentali per evitare che domani siano i mercati, nella miopia che molte

semplicemente per aggiungere ai ringraziamenti già espressi all'Ufficio Parlamentare del Bilancio quelli questa volta ancora più doverosi, sentiti e necessari - al personale e ai funzionari delle Commissioni bilancio e del Servizio del bilancio. È sempre arduo districarsi tra i numeri nei tempi ristretti che in queste occasioni vengono dati al Parlamento. Questa volta - lo abbiamo capito capito tutti - è stato un lavoro ancora più intenso perché ha richiesto un supplemento di indagine. Il lavoro ha potuto svolgersi positivamente e con successo sicuramente grazie al loro supporto e contributo.

intendo cominciare proprio dalla formulazione dei pareri, perché l'oggetto specifico di questa replica riguarda esattamente

Per quanto riguarda le proposte di risoluzione sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, formulerò immediatamente i pareri.

la sua interruzione è opportuna perché mi consente di spiegare qual è la caratteristica della formulazione del giudizio di accettazione

delle caratteristiche fondamentali della manovra di bilancio che l'Esecutivo deve presentare per la sessione di bilancio. Ove il Governo questo come quelli *pro tempore* - si pronunciasse in maniera ambigua, per esempio favorevolmente a un numero rilevante di risoluzioni, ne emergerebbe l'impossibilità di dedurre dal voto del Parlamento l'indicazione esatta circa le caratteristiche e i contorni della manovra di bilancio da presentare per la sessione di bilancio. È per questa ragione che io, pronunciandomi per l'accettazione da parte del Governo della risoluzione n. 2, debbo aggiungere che, tra quelle presentate, ci sono le risoluzioni n. 3 e n. 4

Pronuncio un giudizio politico partitamente su queste due proposte di risoluzione, dopo aver detto chiaramente che quella accettata dal Governo (e che ora è sottoposta all'eventuale iniziativa emendativa) è n. 2, presentata dalla maggioranza. La proposta di risoluzione n. 3 affronta, in particolare, il tema delle politiche verso il Mezzogiorno finalizzate, cioè, ad ottenere un ritmo di crescita del Mezzogiorno più intenso di quello del resto del Paese, così da riprendere la strada della chiusura di questo *gap* che durante la grande recessione, come sappiamo, si è

contenga un'accentuazione ulteriore rispetto a ciò che è contenuto nella risoluzione n. 2 accettata dal Governo. È chiaro che per le ragioni che ho spiegato non posso fare altro che invitare i proponenti al ritiro. Se insistono non avranno un giudizio di accettazione per la ragione di carattere tecnico che ho cercato di far emergere, ma voglio sottolineare che che accetterei, se si trattasse di un ordine del giorno al di fuori di questa procedura, questa indicazione perché nella sostanza contiene impegni che il Governo è disposto ad assumere. In larghissima misura ciò vale anche per la risoluzione n. 4. Ho già spiegato perché il riferimento alla risoluzione n. 2 è esaustivo in questa procedura. È per questa ragione che invito anche i proponenti della proposta di risoluzione n. 4 a ritirarla per non dover formulare su questa implicitamente, per la ragione che ho detto, La valutazione del Governo è la seguente: in premessa sono contenuti valutazioni e giudizi politici di ricostruzione della vicenda politica nazionale e della politica economica nazionale nel corso di questi anni

Come sappiamo, le politiche di contrasto al disagio sociale hanno una componente di sostegno al reddito particolarmente significativa, ma a nostro avviso non si esauriscono nelle operazioni di sostegno al reddito. Ci sono molti interventi sul versante dei servizi alle persone in particolare situazione di disagio sociale che hanno forse un maggiore effetto di sollievo sulle loro condizioni rispetto alle misure di mero sostegno al reddito. Per questa ragione, nello specifico, se si votasse e se il Governo dovesse pronunciarsi su questa proposta di risoluzione, chiederei prima che su questo punto ci fosse una modificazione.

utilizzate, ma fare debito per cose che non servono è quanto di più drammatico ci possa essere, se pensiamo ai nostri cittadini che non riescono ad arrivare a fine mese.

Presidente, le imprese non hanno commesse di lavoro, non hanno soldi per comprare i macchinari, quindi cosa se ne fanno del superammortamento, se non riescono a comprarsi i macchinari? Abbiamo sentito parlare

il primo documento, quello preparatorio della prossima legge di stabilità, da un lato abbiamo una reale curiosità di vedere come si saprà tradurre, in termini concreti, dall'altro oggi non possiamo che rendere all'Assemblea e ai cittadini italiani una grande preoccupazione. Ci sembra

che in questo momento vive il nostro Paese e di quali siano le possibili, reali e forti vie di uscita. Vorrei concentrarmi su un aspetto, che voglio riportare quasi come un virgolettato:

Il rallentamento è da porre in relazione ad un indebolimento della domanda interna, ad una minore dinamica sia dei consumi che degli investimenti,

e consegna al Parlamento la certificazione del proprio fallimento assoluto sul piano delle politiche economiche, perché queste stesse parole erano state messe a supporto di quella nota iniziativa degli 80 euro in busta paga, alla vigilia delle elezioni europee. Tale iniziativa, doveva servire ad accelerare i consumi e quindi, in maniera virtuosa, la produttività, e poi ancora il gettito fiscale. Ma quando si va a discutere del terzo DEF del Governo Renzi non si può più dire «vedremo», «faremo»;

la sopravvivenza del nucleo familiare perché è riuscito ad ottenere un altro prestito da una banca? Quando mai una politica che sia del buon padre di famiglia è orgogliosa di questo e non di poter proporre al proprio nucleo familiare, a chi

In questo DEF voi non tenete conto di ciò che è sotto gli occhi di tutti ed è vissuto in maniera drammatica dai cittadini italiani. Ancora una volta, nella legge di stabilità che si prospetta per l'anno 2017 avrete davanti un Paese profondamente spaccato, diviso,

come rispondete? Con una frase, mi consenta, vice ministro Morando, ipocrita, troppo ipocrita. Lei dice: purtroppo,

una forma invidiosa di un Sud che guarda a un Nord che se la passa meglio: purtroppo, è tutta l'Italia che va male, che non cresce, che non crea occupazione. Ma mi consenta:

i livelli del secondo dopoguerra non può non rendersi conto che ormai gli Stati Uniti e l'Australia sono diventati la meta dei nostri giovani per sbarcare il lunario.

nulla che possa dare il senso di una svolta sul piano economico. Mi è capitato di ascoltare, nella stessa sera, in due programmi diversi, il ministro Delrio dire che la prossima legge di stabilità avrebbe puntato sulle infrastrutture e sugli investimenti infrastrutturali. Poi, a «Porta a Porta», la stessa sera, ho sentito il primo ministro Renzi dire che si sarebbe puntato sulle politiche sociali e sull'aumento delle pensioni minime, e ancora, il giorno successivo,

Voi non avete capito che c'è un tempo per la campagna elettorale, c'è un tempo per fare affermare nelle urne il proprio pensiero, ma c'è un tempo poi del governare. C'è l'etica della responsabilità. Voi dovete farvi la vostra brava campagna elettorale per il vostro stramaledetto «sì» alle riforme che, in maniera raccogliticcia, vi siete votati in Parlamento, ma non potete confondere la campagna elettorale referendaria con l'interesse principale,

di cui ha parlato nel suo intervento il collega Mandelli è un danno oggettivo all'economia. La fiducia è uno degli indicatori fondamentali per la ripresa economica. Il Governo non ha solo il dovere di convincere un Parlamento o la maggioranza dei Parlamenti, rispetto alla propria permanenza a riscaldare le poltrone di Ministri o di governanti; ha il dovere di indicare anche al Paese

porzioni più delicate e indifese della nostra società (mi riferisco alla scuola, ai sei milioni di nuovi poveri che ha il nostro Paese), ma è criminale in quanto si ammazza la speranza delle nuove generazioni. È immorale non riuscire

gli ultimi dati ISTAT, relativi al periodo 2011-2015, mostrano la lunga crisi del Paese. Ma questa tendenza

cambia e archivia le politiche di austerità, dando luogo ad interventi di carattere espansivo che comportano una crescita della domanda interna. L'effetto di fine anno è una riduzione della pressione fiscale di 0,6 punti di PIL, che tuttavia Eurostat contabilizza come aumento di spesa corrente, trattandosi di misure discrezionali non generalizzate. Il *bonus*, sotto forma di fiscalizzazione dell'IRPEF, è infatti garantito solo ai lavoratori dipendenti

sta il fatto che il 2014 si chiude con un leggero incremento del PIL, pari allo 0,2 per cento, chiudendo un biennio negativo. Alla pur limitata svolta ciclica hanno contribuito fattori diversi. La domanda interna, seppur rimasta in territorio negativo con un'ulteriore caduta dello 0,4 mostrato un netto miglioramento rispetto all'anno precedente. L'inversione ciclica determina immediati effetti positivi sulla dinamica della finanza pubblica. L'inversione ciclica, dovuta alla diversa politica economica del Governo, ha condizionato gli sviluppi per l'anno successivo. Se si fosse tornati nel 2015 ad una politica di austerità, i contraccolpi sull'economia reale sarebbero stati devastanti. La carenza di domanda interna avrebbe determinato nuovi e maggiori fallimenti. Nel 2015 invece il PIL cresce dello 0,7 per cento, grazie al contributo della domanda nazionale, che aumenta dell'1 per cento, e delle scorte che, seppur ridimensionate, aumentano dell'0,1 La maggiore crescita migliora decisamente il profilo della finanza pubblica. La spesa corrente, al netto degli interessi, rimane più o meno stazionaria, con un leggero aumento di meno di un miliardo. Le previsioni per il 2016 sono coerenti con il *trend* degli ultimi due anni, anche se non mancano elementi d'incertezza. Secondo la Nota di aggiornamento, il PIL dovrebbe crescere dello 0,8 per cento, grazie soprattutto al forte contributo della domanda interna, L'apporto dell'estero sarebbe invece negativo, per 0,3 punti, mentre le scorte aumentano. L'unico dato certo è dato dalla crescita acquisita alla fine del secondo trimestre, che l'ISTAT valuta nello 0,6 Le incertezze non mancano. Sul piano della finanza pubblica, in attesa che il Ministro dell'economia possa risolvere alcuni dubbi, cerchiamo di giungere ad un giudizio di sintesi di questi primi tre anni del Governo Renzi. La prima cosa da ricordare è che l'inversione del *trend*, rispetto alle precedenti gestioni di Monti e Letta, si è realizzata è realizzata nel rispetto sostanziale delle regole europee, cose, entrambe, non scontate. Si poteva fare di più? Certamente, ma a condizione di non dimenticare che spesso «il meglio è nemico del bene». Non sarebbe, tuttavia, serio non cogliere nel *trend* descritto lacune e contraddizioni, a loro volta riflesso - questo almeno il nostro giudizio - di problemi non risolti innanzitutto sul piano politico. La base parlamentare del Governo è fragile. Le scelte di politica economica sono state osteggiate sia da una parte consistente del partito di maggioranza relativa, sia da quelle opposizioni che hanno scelto la via del nichilismo, piuttosto che il confronto di merito, vale a dire la ricerca di un dialogo che non fosse semplice pregiudizio. Entrambe queste posizioni sono state sconfitte dai numeri che abbiamo illustrato. Pur con mille difficoltà, il Paese è andato avanti, correggendo le precedenti scelte di politica economica. Si è trattato di una politica che non corrisponde alla tradizionale impostazione culturale della sinistra? Forse. Ma in economia vale un vecchio detto del presidente Mao: «Non importa se i gatti siano bianchi o neri; l'importante è che prendano i topi». La politica del Governo non sarà, quindi, una politica di sinistra, comunque è stata una politica efficace, pur nel contesto di una crisi profonda che non riguarda solo l'Italia, ma l'intera Europa. Poteva essere più incisiva se non fosse stata avversata da opposti, per così dire, estremismi. Renzi erede di Berlusconi. Renzi dipinto come il grande imbroglione. La cosa da comprendere è che questo fragile equilibrio non regge più. Ma il dato più evidente è uno ancor più sostanzioso: il mondo sta cambiando e non si va verso il meglio. I prezzi del petrolio, dopo il forte calo dei mesi precedenti, a seguito delle recenti decisioni dell'OPEC, hanno, per lo meno, interrotto la loro rincorsa al ribasso. A fine anno vi sarà un cambiamento della politica monetaria americana, ancora accomodante per via delle prossime elezioni presidenziali. Nel frattempo, il commercio mondiale è crollato. Il suo tasso di crescita, di solito un multiplo della crescita complessiva del PIL, sarà sovrastato da quest'ultimo indicatore, segno del cambiamento intervenuto in tutte le politiche economiche, dove la domanda interna ridiventa elemento traente. Quei grandi volani che hanno sostenuto quel poco di sviluppo in Italia, senza considerare la crisi del sistema bancario, stanno quindi venendo meno. Di fronte a questi scenari occorre un Governo in grado dì operare con il massimo di efficienza, ma questa prospettiva può essere perseguita solo se alla base vi è una maggioranza compatta e maggioranza compatta e coesa, in grado di avere una base programmatica condivisa, che non sia il minimo comune denominatore di opposte visioni. Il mio Gruppo è da tempo consapevole di questa necessità. Ci siamo mossi da tempo lungo questa prospettiva. Spetta ad altri scegliere, nella speranza che, alla fine, la consapevolezza della necessità di perseguire l'interesse nazionale prevalga sulle piccole astuzie del proprio tornaconto individuale. Ballare sulla tolda del Titanic è l'esercizio

il Governo è stato prudente nelle stime riportate, stime che rispetto al Documento di economia e finanza dello scorso aprile sono viste tutte al ribasso. Dobbiamo però tenere presente che i dati programmatici riportati nella Nota risentono degli effetti del «mutato quadro internazionale e del rallentamento della domanda interna». La Nota fissa al 2,4 per cento l'indebitamento netto programmatico delle pubbliche amministrazioni per l'anno corrente (in linea con il dato tendenziale riportato per il 2017, maggiore di 0,4 punti percentuali di PIL rispetto al tendenziale. La richiesta del Governo di autorizzazione a modificare, sino ad un massimo di 0,4 punti di PIL, il tasso di indebitamento netto e quindi il percorso di avvicinamento al pareggio di bilancio è motivata, come abbiamo avuto modo di discutere in Commissione, non solo dai fattori esogeni, che sono quelli che citavo prima, ma anche in relazione ai processi di immigrazione e dalle conseguenze dei recenti eventi sismici che richiedono, ovviamente, ovviamente, interventi straordinari. Peraltro, può essere utile anche per invertire la tendenza al calo della crescita. I dati tendenziali e programmatici riportati nella Nota e confermati ieri dal Ministro richiedono comunque una riflessione. Una riflessione che non va fatta solo sui saldi ma anche, come dice il Governatore della Banca centrale europea Mario Draghi, sulla composizione delle misure di bilancio. In questo senso, le scelte che opererà il Governo saranno determinanti per il futuro. Come sappiamo, gli effetti delle riforme strutturali si vedranno nel tempo ed è quindi necessario proseguire il percorso di consolidamento avviato e al contempo definire politiche di bilancio orientate alla crescita. Per questo riteniamo che il quadro programmatico di finanza pubblica delineato nella Nota, che prevede la disattivazione delle clausole di salvaguardia nel 2017 (pari a ben 15,5 miliardi di euro), scongiurando così l'aumento delle imposte,

della disattivazione di tali clausole e far crescere l'economia del nostro Paese. Così come va portato avanti con più incisività il programma di dismissione e valorizzazione del patrimonio pubblico e di privatizzazione delle partecipazioni societarie. Determinante è puntare anche sugli investimenti pubblici e privati che sono in grado di stimolare la domanda e la crescita della produttività in settori diversificati dell'economia. Per quanto riguarda gli investimenti pubblici, molta importanza assumono quelli volti a mettere in sicurezza il nostro Paese (mi riferisco all'adeguamento antisismico del territorio, al risanamento ambientale e idrogeologico, alla messa in sicurezza dell'edilizia scolastica). In tema di investimenti privati, invece, riteniamo importante stimolarli attraverso misure a favore delle imprese che agevolino l'acquisto di macchinari, delle attrezzature, di beni materiali ed immateriali e misure che favoriscano investimenti in innovazione, ricerca e sviluppo. Condividiamo, quindi, il percorso che è stato illustrato dal Governo in questo senso. Riteniamo poi necessari interventi a favore dei bilanci comunali e degli enti locali. ricordo che con la riforma della legge n. 243 del 2012 si è stabilito che dal 2020 il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa entri nel saldo delle autonomie locali. La stessa legge prevede che sia la prossima legge di bilancio che sia la prossima legge di bilancio a regolare la transizione nei tre anni che ci separano dal 2020, stabilendo la qualità e la quantità della progressiva introduzione nel saldo del Fondo, in modo che risulti compatibile, effettivamente, con gli obiettivi di finanza pubblica. Ci auguriamo, quindi, che tale previsione sia effettivamente contenuta nella nuova legge di bilancio, così come ci auguriamo che siano anche favoriti i processi di fusione e di unione fra le autonomie locali. Inoltre - e si tratta di una questione che ci sta particolarmente a cuore, come ben sa il Vice Ministro auspichiamo che sia attuata una coerente regolazione dei rapporti finanziari tra il Governo, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province Autonome di Trento e di Bolzano,

Questo è un punto che riteniamo strategico, sul quale vigileremo in vista della prossima legge di bilancio con grande attenzione, proprio perché su questo c'è stata un'intesa, che ha una valenza statutaria per le nostre risorse,

di uscita flessibile dal mercato del lavoro e di innalzamento della *no tax area* per i redditi da pensione. Gli interventi delineati su questi argomenti ci sembrano rispecchiare quanto anticipato dai *media*. Certamente troveranno conferma nella prossima legge di bilancio, così come la misura che consente il cumulo gratuito dei periodi contributivi. Determinante è tuttavia anche puntare su una politica fiscale strutturale. In questo senso, auspichiamo che siano previste misure permanenti di riduzione del cuneo fiscale sul lavoro: questo, a nostro parere, è un elemento fondamentale per fare ripartire la crescita nel vero senso della parola. Non vanno poi trascurate le politiche a favore delle famiglie, a sostegno dei carichi familiari e quelle volte a promuovere il diritto allo studio universitario. In questi settori i percorsi delineati sono sicuramente condivisibili. Ben vengano poi le misure volte a prorogare le maggiorazioni degli incentivi in materia di riqualificazione edilizia e per l'efficientamento energetico. Tali incentivi hanno avuto molto successo negli anni scorsi e prorogarle significherà anche dare ossigeno a un settore produttivo che comunque è ancora in sofferenza. Riteniamo poi importante, ai fini della credibilità del nostro Governo di fronte agli investitori europei e del mondo, affrontare il nodo delle banche e del sistema creditizio, cominciando col risolvere l'annosa questione dei crediti deteriorati, che pesano come macigni soprattutto sui bilanci delle banche più piccole. A questo proposito, auspichiamo che siano quanto prima resi pubblici, così come riferito dal Governatore della Banca d'Italia, i dettagli e le analisi dei bilanci degli istituti minori: una trasparenza auspicata auspicata per rassicurare gli investitori e i risparmiatori sullo stato di salute delle banche interessate. Per concludere, merita un cenno anche la politica monetaria: essa dovrebbe essere, a nostro avviso, coordinata meglio con tutte le politiche fiscali dell'Eurozona e mi riferisco anche a quanto discusso questa mattina. A marzo prossimo scadrà il programma di acquisti di obbligazioni governative da parte della Banca Centrale Europea. Se tale programma non verrà esteso si rischiano gravi conseguenze, quali l'aumento degli interessi sul nostro debito e difficoltà per i soggetti interessati ad ottenere prestiti per gli investimenti. Quindi, una politica monetaria espansiva e coordinata può fare la differenza.

Presidente, leggendo e studiando attentamente questa Nota di aggiornamento al DEF e, per la verità, anche sentendo la relazione del senatore Del Barba, mi è venuto in mente che forse si potrebbe coniare un nuovo tipo di valutazione, magari da introdurre attraverso un dispositivo legislativo.

che prima o poi vedremo, come uno strumento di pura propaganda. Il problema è che poi il 4 dicembre arriva, e arrivano anche il 5 e il 6

al costo delle elezioni e della consultazione, ma al costo delle operazioni che sono state messe in atto. Perché si vuole dipingere il Paese come non è. La situazione del nostro Paese è molto problematica, ma il Governo e anche questa Nota di aggiornamento non sembrano accorgersene. Purtroppo, sono cresciute le disuguaglianze, la disoccupazione e la povertà, con un'economia ‑ e questo è il dato drammatico ‑ che non accenna a ripartire. Si ha una ripresa inferiore, molto inferiore a quella degli altri Paesi europei. I numeri della povertà assoluta sono impressionanti, quelli della povertà relativa altrettanto, per non parlare degli 11 milioni di italiani che hanno rinviato o rinunciato alle cure.

è ultima per numero di giovani laureati e quart'ultima per risorse investite nelle università in rapporto al PIL, oltre al fatto che diminuiscono drammaticamente gli iscritti alle università stesse. questa Nota di aggiornamento sia la prova provata del fallimento delle politiche economiche del Governo. L'imbarazzante *iter* - non posso che definirlo così che ha accompagnato l'esame della Nota di aggiornamento in Parlamento - ahimè - sta qui a confermare l'inefficacia delle politiche attuate sinora, altrimenti non si sarebbero nascosti i dati e non si sarebbero utilizzate una serie di furbizie su cui poi tornerò. Tutte le stime contenute, riviste al ribasso già precedentemente, sono state bocciate dalla Banca d'Italia, dalla Corte dei conti e infine dall'Ufficio parlamentare del bilancio, che il vice ministro Morando e anche il presidente della della Commissione bilancio Tonini hanno sempre considerato un po' come il loro gioiello: in tutti questi anni hanno lavorato molto per la costituzione dell'Ufficio parlamentare del bilancio, che doveva essere un organo terzo. Quest'ultimo, con una decisione senza precedenti, ha formulato un esito non positivo del processo di validazione. In tal senso, trovo assolutamente sorprendente, come abbiamo trovato sorprendente ieri sera il ministro Padoan, che peraltro oggi è assente, la pervicace testardaggine con cui il ministro Padoan conferma queste stime, tirando diritto e anche, come abbiamo sentito oggi dalla relazione,

del Governo, che a me sembrano sempre una ripetizione di una sorta di *bonus*, ma di *bonus* in *bonus* finiremo in *malus*. A dimostrazione del livello di irresponsabilità raggiunto dal Governo vorrei stigmatizzare le prime pagine del documento, in cui si attribuisce alla vittoria del «sì» la capacità di far lievitare la crescita economica del nostro Paese nel 2017. Ancora, l'incongruenza delle stime appare evidente anche attraverso le ridicole furbizie

per cento, dal rinvio dell'aumento dell'IVA al 2018, ossia dalla sterilizzazione, ancora per un altro anno, della clausola di salvaguardia. Quindi, il mancato aumento di un'imposta dovuto al suo rinvio viene trasformato dal Governo in una misura di riduzione fiscale connessa alla crescita. Fra l'altro, la politica della riduzione o del contenimento della spesa pubblica per indirizzarne i risparmi verso sgravi fiscali a pioggia in favore delle imprese o per *bonus* fiscali per le famiglie non ha prodotto i risultati sperati.

In questo modo e con questo tipo di impostazione, non solo non si è avviata la ripresa economica, ma non è aumentata la buona occupazione, né è cresciuta la domanda interna. Le politiche di liberalizzazione del mercato del lavoro messe in atto non hanno creato nuovi posti duraturi e dotati di tutela; si è registrato, invece, un aumento del lavoro precario, in particolare dei *voucher*. Riformando il mercato del lavoro si è creato un mercato dei lavoratori sotto ricatto e senza diritti.

Garanzia Giovani, che invece continua a produrre risultati pessimi. Quando arriverà la relazione della Corte dei conti europea, dovremo riparlare della Garanzia Giovani.

lo vediamo - cosa sia esattamente Casa Italia. Sappiamo con certezza che un piano vero di investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio nel nostro Paese non

che si sarebbero dovuti avviare un reale programma di investimenti pubblici, un piano del lavoro, la difesa del *welfare* e il rilancio delle istituzioni.

ma arrivare a un allargamento unilaterale del rapporto - *deficit*-PIL al 3 per cento. È pertanto necessaria una totale inversione di rotta: una manovra triennale complessiva per il lavoro, lo sviluppo, l'innovazione, la ricerca e i diritti sociali di oltre 30 miliardi annui,

lo scorso aprile, del Documento di economia e finanza avevamo registrato la prima vera inversione di tendenza nel nostro Paese dopo la crisi economica degli ultimi anni. Nel 2015 il prodotto interno lordo è aumentato, la disoccupazione e le tasse sono diminuite e le riforme strutturali per il Paese erano in corso di approvazione e di attuazione. In altre parole, l'Italia si è rimessa in moto ed è tornata finalmente a crescere. Ciò che è stato fatto finora ha rappresentato una fondamentale inversione di tendenza, ma allo stesso tempo non può essere che il primo di una serie di punti positivi per una piena e consolidata ripresa. Siamo soddisfatti delle riforme fin qui attuate, dei provvedimenti di rilancio dell'occupazione e degli investimenti. Ma tutto ciò non può che essere uno stimolo affinché Parlamento e Governo continuino sul percorso riformatore. L'operato della maggioranza, sin dal suo inizio, ha perseguito una strategia orientata al rilancio degli investimenti, pubblici e privati e, in modo particolare, al sostegno dei consumi interni attraverso l'aumento del reddito disponibile delle famiglie e la riduzione della pressione fiscale, scesa dal 43,6 del 2013 al 42,1 del 2016. Questi fattori chiave, assieme all'ambizioso programma pluriennale di riforme strutturali, stanno contribuendo a migliorare la competitività del sistema produttivo. Lungi dal sentirci appagati, siamo consapevoli del fatto che l'anno passato deve costituire la base per uno sviluppo più solido e strutturato che coinvolga tutti i settori del Paese. La maggioranza e il Governo sono ben consci che gli ostacoli da superare per arrivare ad una piena ripresa sono ancora molteplici e radicati da troppo tempo nel nostro sistema Paese. Non a caso, il ritmo della ripresa è rallentato oltre che dalla durezza della doppia e profonda recessione che ha caratterizzato il periodo 2009-2013, anche dal peggioramento delle prospettive di crescita a livello internazionale, dall'invecchiamento demografico, dal ridotto tasso di innovazione, dall'incertezza sulla *governance* dell'area europea e dai persistenti squilibri macroeconomici, che si associano a tassi di interesse e d'inflazione su su livelli storicamente assai contenuti e prossimi allo zero. D'altra parte, nel delicato equilibrio tra necessaria ristrutturazione dei conti pubblici e stimolo alla crescita, non possiamo trascurare la parte propulsiva della nota di aggiornamento al DEF. L'aumento degli investimenti in infrastrutture permetterà sicuramente uno stimolo della produttività in numerosi settori dell'economia. In questo ambito, l'Italia è il secondo Paese in Europa per l'utilizzo dei fondi del Il tema degli investimenti infrastrutturali dovrà necessariamente includere la costruzione del ponte sullo stretto di Messina, che rappresenterà il culmine di un lungo processo volto a concretizzare l'impegno preso dal Governo in merito al completo superamento del *gap* infrastrutturale che separa il Sud dal resto del nostro Paese. non solo consentirà il completamento del corridoio Nord-Sud a livello europeo, ma consentirà maggiori e più facili flussi di persone, merci tra la Sicilia e l'Italia, con stimoli economici di estremo rilievo. Con la nota in esame, il Governo ha indicato una maggiore gradualità nel raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, indicando un indebitamento netto pari al 2 per cento del PIL per il 2017, superiore di 0,2 punti percentuali rispetto a quanto previsto ad aprile nel DEF,

Queste stime al ribasso sono state determinate da alcuni eventi eccezionali, quali gli eventi calamitosi che hanno colpito lo scorso agosto le popolazioni del Centro Italia. A tal proposito, come già sottolineato dalla mozione approvata in Senato qualche settimana fa, chiediamo rigore e lungimiranza nel delineare gli strumenti, anche eccezionali, per mettere in sicurezza il territorio, il patrimonio abitativo e le infrastrutture scolastiche, nonché il risanamento ambientale e idrogeologico. Per il risanamento del patrimonio abitativo, nello specifico, riteniamo opportuno prorogare ulteriormente le maggiorazioni delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni e l'efficientamento energetico, rendendole effettivamente fruibili anche per i grandi condomini, al fine di tutelare l'ambiente, consentire la ripresa dell'occupazione nell'edilizia e favorire l'innovazione tecnologica nel settore.

la conferma di agevolazioni quali il superammortamento e la sua declinazione in base al tipo di investimento in beni strumentali, nonché la previsione di ulteriori agevolazioni in favore degli investimenti in innovazione, ricerca e sviluppo, il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e gli interventi volti a favorire la crescita dimensionale e l'internazionalizzazione delle imprese. Il sistema produttivo dovrà essere sostenuto, inoltre, attraverso un rafforzamento della detassazione dei premi di produttività, nonché mediante lo sviluppo delle piccole e medie imprese, da garantire attraverso un medesimo livello di tassazione per le diverse forme giuridiche in cui l'impresa viene ad organizzarsi. L'azione di rilancio delle aree sottoutilizzate e la riduzione delle disparità regionali si deve realizzare assicurando la piena attuazione del *masterplan* per il Mezzogiorno e definendo le azioni strategiche specifiche per ogni area territoriale interessata. In merito al sistema pensionistico, ben vengano le misure volte a garantire flessibilità in uscita, a patto che non vi siano aggravi spropositati per i beneficiari: il cumulo gratuito dei periodi contributivi, le forme di sostegno all'uscita flessibile dal mercato del lavoro, l'aumento dei trattamenti pensionistici di importo basso, le azioni in favore dei lavoratori precoci e usuranti sono tutte misure che devono essere tarate nell'ottica di un'entrata nel mondo del lavoro dei giovani. Per ultimo, ma non per importanza, cito il capitolo relativo alla famiglia. Auspico che la prossima legge di bilancio contenga un capitolo nutrito di misure a sostegno del nucleo familiare, che garantisca agevolazioni, legati all'ISEE, in favore dei nuclei familiari, per le spese legate all'istruzione, alle attività sportive e alla crescita dei figli. Vorrei esprimere, in conclusione, l'apprezzamento personale e del Gruppo a cui appartengo, per l'orizzonte futuro delineato in questa Nota di aggiornamento, caratterizzata da coraggio e prudenza, determinazione e consapevolezza, innovazione e ponderatezza.

Non volevo votarla, perché onestamente non so nemmeno che cosa stiamo votando. Abbiamo esaminato una Nota d'aggiornamento al DEF, che non è stata validata dall' Ufficio parlamentare di bilancio, per quanto possa ritenerlo piuttosto

Ho sentito proprio una nota di imbarazzo ad ascoltarlo, in qualità di parlamentare che avrebbe dovuto avere delle giustificazioni e delle ragioni, che poggiassero su modelli concreti e criteri oggettivi, che invece non ci sono.

ma siccome sta facendo nuovo *deficit* e riesce a bloccare se stesso per quest'anno, soltanto per questa ragione si crescerà dello 0,3

quando avete apposto questa clausola di salvaguardia avete minimamente considerato gli effetti recessivi. Avete alzato l'aliquota IVA così, con leggerezza. Comunque ho fatto un'altra domanda al ministro Padoan: secondo i deflattori al consumo, guardando sia la parte tendenziale che quella programmatica e facendo il paragone tra il 2017 e il 2018,

tutto il resto è traslato negli anni avvenire. Se devo credere che riuscirà a bloccare 20 miliardi di nuove tasse a partire dal 2018,

Questo perché la nuova flessibilità non serve a fare gli investimenti; essa proverrà da un'Unione europea altamente politicizzata che, per fermare il Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo e gli altri movimenti nel resto d'Europa, darà

che gli darà finalmente la finta abolizione del Senato, con il finto risparmio del miliardo di euro che aveva promesso. In realtà il nostro bilancio si mantiene su un solo pilastro, cioè cioè sull'abbattimento del costo degli interessi passivi sul debito, che però non è opera di Renzi, ma della politica espansiva di Draghi, che però finirà. E allora altro che pensare al famoso *spread* di quando c'era Berlusconi! Presentando un documento di questo tipo i mercati impazziscono, a meno che non ci sia un Governo serio e autorevole che, anziché giocare con i *bonus*, i *tweet* e alla *PlayStation,* parla dei problemi del Paese e vuole finalmente fare quegli investimenti che ormai suggeriscono tutte le istituzioni nel mondo. Non siamo solo noi a essere arrivati qui nel 2013 con questa fissa:

È curioso vedere che nei prossimi anni le amministrazioni centrali non faranno altro che aumentare l'asticella del debito pubblico, mentre quelle che concorrono a risanare la finanza pubblica sono le amministrazioni locali, cioè Regioni e Comuni. e Comuni. E sappiamo che già dall'anno prossimo scattano quattro miliardi di tagli alla sanità. State giocando anche con il Fondo sanitario nazionale, perché non lo aumenterete. Qui dentro volete mettere una rappresentanza territoriale delle Regioni, quando in

lo aumentate, allora lo tagliate. E tagliate alle amministrazioni locali che hanno il primo approccio con i cittadini. Questo fate, mantenendo le mani libere alle amministrazioni centrali per continuare a dare i contentini a destra e a manca e per mantenersi a galla. a galla. Io, onestamente, avrei preferito anche non votare questo DEF, perché è un documento vuoto in cui è sancito l'ennesimo fallimento del Governo Renzi e, purtroppo, anche la perdita di credibilità del ministro Padoan, che doveva essere soltanto un tecnico ma si è rivelato rivelato essere un soldatino, che sta facendo soltanto la politica di Renzi, arrancando e andandogli dietro. Signor vice ministro Morando, io non posso credere che lei non sappia che, in realtà, noi ci manteniamo a galla soltanto per la diminuzione degli interessi passivi tutta la politica economica di questo Governo è fallimentare. Noi cresciamo meno degli altri, altro che locomotiva europea. Noi abbiamo un livello di disoccupazione, rispetto alla media europea, più alto rispetto a quando è arrivato Renzi. È fallito il *jobs act* ed è fallita la decontribuzione, con quell'imbroglio per cui state aumentando cui state aumentando il cuneo fiscale di un miliardo a carico delle imprese artigiane. E vi mantenete con la finta lotta all'evasione, fatta dallo *split payment* che ha messo in ginocchio le nostre aziende che lavorano con la pubblica amministrazione.

votare contro questo DEF e contro la mozione che ne promuove l'approvazione, più che semplice, è quasi dovuto. Questo si costruisce sulla base di un presupposto che tante volte ho sentito pronunciare come bestemmia da parte di colleghi, anche autorevolissimi, della Questo DEF si costruisce su un *deficit* programmatico che peggiora quello tendenziale. Ciò significa che, programmaticamente, l'azione del Governo peggiora i conti pubblici.

per forza si traduce negli anni successivi in aumento del debito. Ma il Governo dice che, programmaticamente, si peggiorano i conti pubblici. E lo fa in un altro contesto che suonava bestemmia anni fa: in un contesto che vede il peggioramento, da parte di questo Governo, dell'avanzo primario.

i tassi di interesse sono scesi al minimo di sempre. Ora, è chiaro che i due concetti sono profondamente contraddittori. Quante volte ho sentito dire che quando i tassi di interesse scendono si aumenta l'avanzo primario, così poi si possono fare gli investimenti! Come si dice in Italia - mi si scusi per la mia rozzezza - predicano bene e razzolano non male, ma malissimo, con questi due presupposti.

il Governo sostiene questo. Premetto che il Governo, sulla base storica, sa che ha sbagliato tutte le previsioni negli anni precedenti per difetto, non è che un Governo aumenta la manovra perché, basandosi sulla serie storica, ha visto che le sue previsioni miglioravano. Nel Nel 2013 il DEF per il 2014 prevedeva un tasso di crescita dell'1,3 per poi finire allo 0,1. Nel 2014 prevedeva per il 2015 un tasso dell'1,3 per poi finire allo 0,7. Già per il 2016 prevedeva l'1,4; poi DEF 2015 prevedeva addirittura l'1,6. Adesso, come dice il Presidente del Consiglio, siamo allo "zero virgola". Quindi, la base storica deve autorizzare a tenersi cauti, prudenti; e invece no. Il Governo dice: nonostante tutto - lo vedremo alla fine - prevedo l'uno per cento. Quindi, siamo nell'ambito di una opinabilità molto elevata, che dunque conferisce a quel dato una probabilità molto vicina allo zero.

pari a una cifra tendente allo zero perché è straordinario pensare come qualcosa che non si è avverato, l'aumento dell'IVA, è stato incorporato dalla signora che compra ogni giorno i beni, sapeva che c'era questa manovra della clausola di salvaguardia; pertanto, siccome l'abbiamo tolta, lei comprerà di più. Non è così. So perfettamente che noi facciamo i conti su tendenziali e saldi, ciò che abbiamo incorporato ma, a mio avviso, quando si parla di impatto sulla crescita, si parla di impatti sull'economia reale, e quella eliminazione delle clausole, cui il Governo annette il maggior impatto sulla crescita, per me è vicino allo zero.

La traduco (mi si scuserà ma, a pensar bene, come è noto, si fa peccato veniale ma non si sbaglia quasi mai): il Governo dice: siccome con il due per cento non raggiungo l'uno, arriviamo al 2,4, così forse lo raggiungo. Quindi il 2 è chiaramente una cifra che un sociologo che piace molto - credo che

l'Ufficio parlamentare di bilancio. E qui pongo al Parlamento una questione: sul piano giuridico è chiaro che il Governo ha ragione: la sanzione che pone allo sfasamento tra previsioni del Governo e previsioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio la legge di bilancio è che il Governo deve venire a motivare se intende confermare la sua previsione oppure no. Il Governo è venuto e l'ha confermato. Questo, nei rapporti tra Governo e Ufficio parlamentare di bilancio, è corretto. Ma noi in Parlamento che facciamo? L'Ufficio parlamentare di bilancio è l'Ufficio che stima per il Parlamento, nei confronti del Governo, i parametri che deve stimare. Qui c'è una differenza significativa, perché il Governo è andato sopra tutti i parametri di previsione. Il Governo conferma e noi Parlamento non diciamo niente;

a fronte di questo squilibrio (che sul piano giuridico è assolutamente compatibile, ma non sul piano politico), non possa che prevedere al più presto un'iniziativa di sfiducia nei confronti del Governo,

Signor Presidente, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi,

ha risentito in questo difficile 2016 di un rallentamento a livello internazionale molto vistoso. Lo approviamo per sostenere con forza la previsione di crescita dell'uno per cento, che al tempo stesso rappresenta un obiettivo ambizioso e un parametro credibile, attraverso una forte e convinta azione di sostegno a questa crescita. Su questo punto, su cui molti interventi si sono soffermati, vorrei aggiungere che questo obiettivo,

è stato prezioso il lavoro dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che ha permesso, con le sue obiezioni, di approfondire molto seriamente con il Ministro le politiche, le modalità e le motivazioni di questo obiettivo di crescita. Quindi possiamo dire che adesso, dopo queste riflessioni, questo obiettivo rappresenta sicuramente un obiettivo cui tendere, ma anche un obiettivo che è sostanziato da importanti e significative politiche che lo accompagneranno, che sono previste nella Nota di aggiornamento al DEF e che saranno ancora più fortemente esplicitate nella politica di bilancio. A questo proposito non mi voglio sottrarre al fatto che nelle due risoluzioni che presentiamo autorizziamo il Governo a chiedere fino allo 0,4

somma dei due ragionamenti che abbiamo fatto approfonditamente in Commissione - cioè politiche concrete a sostegno dell'obiettivo dell'uno per cento

almeno su questo, abbiamo la testa alta di non dire inesattezze gravi, anche moralmente censurabili

al DEF e la legge bilancio cercano di tenere insieme anche un altro elemento (su cui mi posso dilungare poco, lasciando agli atti il sostegno alla crescita, agli investimenti, all'innovazione, alla ricerca con un piano articolato e serio di tutela sociale, basato sul sostegno al lavoro, sulla lotta alla lotta alla povertà e sul sostegno alla famiglia, affrontando coraggiosamente il tema della previdenza, che da molte parti in questi anni è stato sollecitato e che adesso viene concretamente affrontato. Su questi punti, assieme ad altri, io credo che dobbiamo avere la capacità di dire - e per questo motivo votiamo convintamente a favore delle nostre risoluzioni del DEF - che l'insieme di questi interventi non configura un Paese che vuole guardare indietro, che non crede a quello che può fare, ma un Paese che costruisce testardamente anche la coesione tra le generazioni, tra i giovani e gli anziani perché crede che si possa costruire un di coesione, di crescita, di maggiore sviluppo e di maggiore benessere per tutti. *(Vivi

Procediamo alla votazione della Proposta di risoluzione alla relazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012. Avverto che per tale deliberazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. Pertanto, la votazione della proposta di risoluzione avrà luogo mediante procedimento elettronico con scrutinio simultaneo.

sintesi ampliata di tutte le promesse che sta facendo il Presidente del Consiglio per poter avere il «sì» sulla riforma costituzionale: disattivare nella prossima manovra di bilancio le clausole di salvaguardia, interventi di adeguamento antisismico, il super ammortamento (che mi sfugge), rafforzare la detassazione, le misure per il Trentino-Alto Adige, il *masterplan* per il Mezzogiorno, la pensione, la povertà, i carichi familiari, il fondo sanitario, tutto lo scibile umano. Ovviamente la risoluzione non contiene nulla se non il primo punto che io intendo sostituire con il mio emendamento. Com'è sintetizzabile il primo punto? In pratica impegna il Governo a sforare tutti i conti pubblici e quindi a mandare a quel Paese il bilancio. Chiedo quindi che il Governo si impegni a rendere le stime fornite compatibili con le osservazioni dell'UPB che dovrà provvedere alla conseguente successiva validazione dei dati forniti, come richiesto dalla normativa europea e nazionale, al fine di assicurare il pieno rispetto di tutti i parametri di costituzionalità.

Ricordo a me stesso il 1° comma dell'articolo 117 della Costituzione, che non ci piace e avrei già abrogato o sostituito, ma purtroppo c'è e ci sarà anche se dovesse essere approvata la futura Costituzione, «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario» (che è quello che io francamente avrei soppresso).

siano validate da un'istituzione nazionale indipendente, ovvero l'Ufficio parlamentare di bilancio.

tra lo stesso e il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2014. Presidente, se la normativa e i vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea hanno un senso, visto che c'è un regolamento che rientra in questi vincoli, che è previsto dalla Costituzione, visto che l'UPB è stato istituito con un legge rafforzata (quindi non basta una semplice decisione del Parlamento, ma viene viene richiesta la maggioranza assoluta), con il mio emendamento chiedo: caro Governo, rendi compatibili le tue stime in modo tale che possano essere validate dall'Ufficio parlamentare del bilancio. Se non si vuole neanche questo, si dice già che non si intendono rispettare le richieste e le osservazioni che l'Ufficio ha formulato e quindi si intende sforare i conti pubblici e fare una cosa incostituzionale. Poi sono certo che, essendo la "ciccia" il primo punto degli impegni, nessuno potrà votare sì all'emendamento, ma voglio con questo voto che il Parlamento certifichi l'incostituzionalità

finanze*. Signor Presidente, la proposta è simpatica. Naturalmente il senatore Calderoli ha proposto di sostituire nella risoluzione l'unico capoverso che rende questa risoluzione quella prevista dai nostri regolamenti e dalle norme, perché il Governo, approvata questa risoluzione dal Parlamento, possa predisporre la legge di bilancio. a questa proposta, il Governo non saprebbe quali sono i confini dal punto di vista finanziario e programmatico della legge di bilancio. Il Governo è dunque contrario

settant'anni esatti dal 12 ottobre 1946, quando il Consiglio dei ministri con Alcide De Gasperi decise che quello dovesse essere l'inno nazionale, seppur ancora provvisoriamente. Quindi stiamo attendendo

settant'anni della Repubblica meritino di vedere finalmente una decisione definitiva su questo inno. Ci sono naturalmente dei motivi storici, ma va riconosciuto a Goffredo Mameli e a Michele Novaro che «Fratelli d'Italia», se è arrivato fin qui (l'anno prossimo saranno centosettant'anni dalla sua composizione), evidentemente è perché si è caricato di un significato ed è un simbolo e una citazione di tutto il nostro popolo e del nostro Paese. la proposta c'è e credo che ci sia anche la volontà, in questo settantesimo anniversario della Repubblica, di poter dedicare